senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del senatore Stefano Zuccherini, uomo di vivace intelligenza, forte carattere e grande generosità d'animo. Storico dirigente della FIOM-CGIL umbra e nazionale, Stefano Zuccherini è stato per molti anni la voce più rappresentativa del Movimento operaio, per il quale non ha mai smesso di battersi con instancabile determinazione. La sua esperienza nella politica e nelle Istituzioni era iniziata nel 1993 con l'ingresso nel partito di Rifondazione Comunista e la successiva elezione al Consiglio regionale dell'Umbria, un'esperienza che Stefano Zuccherini ha vissuto con passione, dedizione e coerenza di pensiero. La stessa passione lo avrebbe portato in pochi anni ai vertici della segreteria nazionale del partito e lo ha reso una delle sue figure più autorevoli. autorevolezza derivava dall'orgoglio con cui Stefano Zuccherini ha sempre difeso le proprie idee, ma anche la sua libertà di pensiero, e con cui ha vissuto l'impegno politico, quella di un uomo che credeva nel dialogo come valore cardine della democrazia e che guardava al confronto come strumento critico per costruire e risolvere. Si tratta di una genuinità di valori e una ricchezza morale che Stefano Zuccherini portò con sé in quest'Aula come senatore nella XV legislatura, nel corso della quale fu anche vicepresidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, oltre che componente della Giunta delle elezioni e del Comitato per i procedimenti di accusa, incarichi che seppe interpretare con rigore e profondo rispetto per l'Istituzione parlamentare. Con Stefano Zuccherini ci lascia un politico di cuore e di coraggio, un attento lettore delle dinamiche sociali e un sensibile interprete dei diritti dei più deboli, un uomo che ha dedicato tutta la vita alla difesa del lavoro, collegamento fondamentale tra destini individuali e collettivi, come lo ebbe a definire proprio in quest'Aula, nella convinzione che nessuna forma di protezione sociale può compensare la menomazione di diritti di cittadinanza dovuta all'assenza di lavoro o prodotta dalla precarietà. Tale visione oggi, nel pieno della crisi economica e sociale prodotta dalla pandemia, è un'esortazione a non dimenticare che la vera via della rinascita di un'Italia così drammaticamente ferita è quella che inizia dalla tutela concreta di ogni lavoro. In ricordo del senatore Stefano Zuccherini invito pertanto l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

5 marzo 2021, n. 25, all'esame dell'Assemblea per la conversione in legge, reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali: le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; le elezioni amministrative, a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021; infine, le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a Statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verifichino le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Con una modifica introdotta in Commissione affari costituzionali è stato disposto il rinvio, però, anche delle elezioni degli organi delle Città metropolitane, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021, in luogo dei primi sei mesi dell'anno 2021, come già previsto: sono identici gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2). Nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì aggiunto l'articolo 1-*bis*, volto a introdurre una procedura semplificata per la designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021: emendamento 1.0.1 (testo 3). L'articolo 2, invece, prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature sia ridotto a un terzo. Durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti. In particolare si prevede che, limitatamente all'anno 2021, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla. Si dispone altresì che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto (emendamento 2.5). L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate: domenica (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì (dalle ore 7 alle ore 15). Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che, nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per Camera e Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative. Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si dispone inoltre che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e, poi, a quelle circoscrizionali. che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Un ulteriore intervento emendativo della Commissione ha introdotto la previsione, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 (e solo per esse), dell'apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine per la pubblicazione del certificato dei candidati (emendamento 3.0.100 (testo 4)). (testo 4)). La Commissione ha anche approvato due identici emendamenti volti a fissare al 31 ottobre 2021 il termine entro cui devono concludersi le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,

Inoltre, sono stati accolti alcuni ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti. Segnalo, in particolare, un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale (argomento, questo, sensibilizzato sensibilizzato da molte parti d'Italia). Segnalo altresì un altro ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza, con effetto retroattivo, dei permessi riconosciuti dai sindaci in occasione dell'emergenza epidemiologica.

relativamente alla produzione della documentazione richiesta per le candidature.

Signor Presidente, prendo spunto dal provvedimento in esame, che naturalmente credo non possa che vederci

relativa alla dignità politica ed economica degli amministratori locali. Non era questo il provvedimento in cui potevamo inserire tale tema, ma in tutti questi anni abbiamo avuto uno sguardo troppo disattento alla dignità politica politica ed economica degli amministratori locali. Penso ai consiglieri provinciali delle Città metropolitane, che svolgono il loro lavoro a titolo gratuito, penso alle indennità troppo basse

le Province e le Città metropolitane dalla Costituzione. Sono passati quasi cinque anni e dovremmo riprendere in considerazione la questione

deleterio e quindi chiedo che il Parlamento e le Commissioni competenti prendano in mano le tante proposte di legge che ci sono e le portino a compimento. L'ultimo tema dell'estensione della possibilità del terzo mandato per i Comuni sotto i 15.000 abitanti come abbiamo fatto per i Comuni sotto i 3.000 abitanti.

ricominciamo a discutere di enti di area vasta quali Province e Città metropolitane elette direttamente dai cittadini e poniamoci anche il problema del terzo mandato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghi, abbiamo cercato di dare il nostro contributo fattivo a questo provvedimento proprio puntando sulle problematiche degli enti locali di cui il senatore Astorre ha parlato poc'anzi. Abbiamo cercato di far presente quali sono i problemi più urgenti urgenti che stanno affrontando i nostri enti locali, in particolare i più piccoli, anche se ovviamente non è questo il provvedimento per risolvere le tantissime problematiche

un fallimento della classe politica di questo Paese, non dei Comuni. Infatti, abbassare il *quorum* in caso di lista unica significa che ci sono sempre più amministrazioni in cui non c'è gente che vuole candidarsi come sindaco, come consigliere, come assessore. Chiedere di fare il terzo mandato anche nei Comuni con più di 3.000 abitanti o addirittura togliere il limite di mandato nei Comuni con meno di 3.000 abitanti, come noi chiediamo perché ci sono dei problemi contingenti (io da sindaco di un piccolo Comune sotto i 3.000 abitanti sono al terzo mandato e lo so), è comunque un fallimento, perché significa che non c'è ricambio della classe dirigente, di chi governa un territorio. Dobbiamo quindi farci delle domande. Sembra che l'arco costituzionale trasversalmente sia concorde - ne abbiamo parlato anche in Commissione - sul fatto che bisogna finalmente affrontare tutti i problemi dei piccoli Comuni. Ne abbiamo parlato con

ai cittadini la voglia di candidarsi, di lavorare per il proprio paese, per la propria cittadinanza. Se non lo fanno, non è per disinteresse, ma perché fare il sindaco comporta troppe responsabilità

se in inverno c'è la neve e non viene pulita entro due ore si chiama il sindaco; se in estate ci sono allagamenti per le strade, è colpa del sindaco che non ha pulito le caditoie; se in autunno c'è il vento o in primavera succede qualche danno dovuto a calamità naturali,

dell'ufficio tecnico, si ritrova a esser ritenuto responsabile in quanto ha il potere di controllo dell'ente. La stessa cosa capita ai sindaci dei piccoli Comuni, vedono cadere un masso da una montagna (magari nei Comuni montani), e hanno la responsabilità anche in caso di incidente o ancora peggio della morte di qualcuno. Capite bene che fare il sindaco in queste condizioni, oltretutto adesso in piena pandemia, è come vivere con una spada di Damocle sulla testa. Il sindaco non può essere responsabile di cose che non gli competono e non dovrebbe neanche essere responsabile di settori del Comune visto che spesso non ha né gli studi, né le competenze professionali per poterlo fare; eppure deve farlo. Dobbiamo trovare un modo per risolvere questi problemi, per ridare dignità ai sindaci. In questo anno non avete visto proteste nelle piazze e nelle strade da parte dei sindaci, anche se

Mi auguro, visto che abbiamo una maggioranza trasversale e siamo tutti d'accordo sul fatto che i sindaci - in particolare quelli dei piccoli Comuni che, vi ricordo, rappresentano il 70 per cento dei Comuni italiani hanno bisogno di essere aiutati, che si smetta di parlarne e si cominci a lavorare seriamente per riformare gli enti locali, smettendo di parlare di norme imposte, di fusioni e di tagli. che sono i sindaci i primi che sanno risparmiare dove c'è da risparmiare e sanno collaborare con i propri colleghi e con i Comuni vicini quando è utile per la propria cittadinanza. Bisogna smettere di imporre norme che, nel tempo, non sono servite assolutamente a niente.

il problema di fare la spesa e in isolamento totale. Abbiamo ancora uno stile di vita che è da preservare e da valorizzare grazie ai nostri spazi e ai nostri servizi che forniamo ai cittadini. Scusate se

tanta gente, come notate, appena può scappa, legalmente o meno, nelle seconde case di montagna, di campagna o di mare perché vivere in *lockdown* in un Comune di campagna e vivere in città non è esattamente la stessa cosa.

Abbiamo però il problema di raggiungere le scuole superiori perché non ci sono i mezzi adeguati per raggiungere i Comuni che hanno le scuole. Se ne potrebbe parlare veramente all'infinito. È bello avere dei buoni propositi, mi auguro

adeguati per garantire una vita dignitosa ai propri cittadini.

sottolineare l'aspetto che è stato messo in luce dalla collega Pirovano e cioè che il tema del rinvio

in realtà mette in luce una serie di emergenze del nostro Paese che hanno a che fare soprattutto con i Comuni minori, con i piccoli Comuni. Ricordo, tra l'altro, come abbiamo

che, talvolta, sia persino complicato poter eleggere un sindaco e un consiglio comunale. Ci sono addirittura casi nei quali

e un consiglio comunale, evitando di lasciare quel Comune senza guida, con un commissario prefettizio. Le problematiche proseguono: è chiaro che tutto il tema delle elezioni comunali ha a che fare con una risistemazione del quadro nostro Paese, che necessita di un "tagliando" e di una rivisitazione complessiva. Ad esempio, che nei Comuni minori si possa dare la possibilità

diventa difficile trovare persone disponibili a candidarsi a sindaco, per prestare il proprio tempo, le proprie energie

è miglior *testimonial* di chi ha svolto e svolge il ruolo di sindaco ed è costretto ad arrabattarsi, per fare in modo che

presentazione delle liste, facendo in modo che diventi semplice e non difficile presentare le liste per le elezioni comunali. Dobbiamo coinvolgere convincere i cittadini a prendere parte alla vita pubblica del nostro Paese, anche al livello del proprio Comune e, perché ciò accada, non dobbiamo complicare, ma semplificare il quadro normativo per la presentazione delle liste. Credo che lo

e quindi so bene cosa significa affrontare il tema delle elezioni locali e cosa significa non solo andare a chiedere il voto di preferenza, ma soprattutto Non sto andando fuori tema, cari colleghi, perché il tema dello spostamento delle elezioni comunali, collegato a un'emergenza pandemica quale quella che sta vivendo in modo patologico il nostro Paese, ci mette nelle condizioni di fare e questo è un fatto positivo - su una questione che merita un approfondimento. Si tratta del coinvolgimento delle persone alla vita pubblica, alla politica, in una fase nella quale dobbiamo riconquistare l'amore per la politica: dobbiamo convincere, far capire a tutti i cittadini che fare politica

introduce di fatto un tema che merita di essere approfondito, e cioè quello dell'amore per la politica in una fase nella quale tutti i cittadini devono riconquistare fiducia nei suoi che, purtroppo, invece, è andata via via scemando. Questo è compito nostro, cari colleghi: far tornare la fiducia nei cittadini, soprattutto in un periodo nel quale

Per questa ragione, ho colto questa opportunità per ricordare a ciascuno di noi il compito, la missione che dobbiamo svolgere: dare una dare una buona amministrazione al nostro Paese, al nostro Stato, pensando già alle riaperture, alla capacità di produrre fiducia verso un futuro migliore, in un momento nel quale le forze politiche in campo hanno fatto tutte un passettino indietro per guardare avanti con fiducia e unire il Paese per una prospettiva diversa.

dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge gli emendamenti 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 e 3.0.19. 3.0.19. Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis* e gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2. I colleghi vedranno dal fascicolo che alcuni sono stati anche ritirati e, quindi, il problema è

formulo un invito al ritiro, ricordando che è stato approvato un ordine del giorno in Commissione, come giustamente mi è stato ricordato.

al testo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nonché con le tempistiche necessarie all'organizzazione e al relativo approvvigionamento, l'opportunità di adottare iniziative volte alla sostituzione delle attuali urne elettorali con altre di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse». Esprimo parere contrario sul secondo e sul terzo impegno

gli ordini del giorno approvati in Commissione,

per la rielezione del rettore e di tutto il collegio. Il termine del 31 ottobre, indicato come proroga ideale, sicuramente non risolve il problema per quei pochi atenei che,

il decreto che andiamo a convertire oggi fa parte di tutta quella serie di provvedimenti utili a prendere atto del permanere di una situazione pesante dal punto di vista dell'emergenza epidemiologica, che impone comunque delle variazioni per quanto riguarda la tempistica - in questo caso delle elezioni - in altri momenti diversi della vita quotidiana. Quando approviamo provvedimenti di questa natura, il pensiero va sicuramente alla riconquista di una normalità che ancora appare lontana, ma che deve essere il tratto dominante della nostra azione di parlamentari, ma soprattutto dell'azione quotidiana del Governo.

che insieme a tutte le misure di contenimento può veramente determinare la svolta per il Paese e far sì che i provvedimenti che andiamo ad approvare oggi siano qualcosa da dimenticare in fretta. fretta. Speriamo che in questo caso il rinvio delle elezioni, che non è sicuramente il tema che hanno in mente gli italiani, sia uno degli ultimi provvedimenti che mettiamo in campo per rinviare qualcosa e per far fronte al permanere di un'emergenza comunque alta in termini di contagio e purtroppo di decessi, che sono ancora molto alti e lasciano il Paese in un clima mesto e di dolore. Il provvedimento in esame sostanzialmente - come abbiamo sentito già negli interventi precedenti e dalla relazione del relatore - rinvia la data del turno elettorale ordinario che ci sarebbe stato tra aprile e giugno per quanto riguarda le elezioni amministrative,

sciolti per altri motivi, per dimissioni dei sindaci, per impedimento permanente, per il venir meno della maggioranza nei Consigli comunali; insomma per tutte quelle vicende che hanno determinato l'interruzione della vita di alcuni Consigli comunali e quindi la decadenza dei sindaci. In pratica, si sposta il turno elettorale nel periodo che va dal 15 settembre al 15 ottobre, per consentire lo svolgimento delle elezioni in condizioni di sicurezza, chiaramente con un occhio di riguardo nei confronti dei cittadini che si recano alle urne, nonché per consentire a chi deve lavorare in quel contesto - prefetture e personale degli enti locali - di poterlo fare in una condizione di maggiore sicurezza. A settembre-ottobre avremo sicuramente un quadro migliore dal punto di vista della tenuta del Paese, perché avremo sicuramente un livello molto alto di vaccinazione e, quindi, di immunizzazione. Il provvedimento al nostro esame - nella dichiarazione di voto è giusto fare delle considerazioni di carattere politico - è stato migliorato con un occhio di riguardo alla vita delle amministrazioni comunali. Credo sia stato questo - come già evidenziato in molti interventi - un punto importante, con tutti gli emendamenti approvati, tesi a ridurre gli adempimenti e a dare dignità - come prima è stato detto - a situazioni in cui vengono presentate, ad esempio, singole liste per le elezioni comunali,

Sono stati introdotti elementi migliorativi per la vita dei sindaci, di fatto eliminando le sanzioni per una presentazione tardiva della relazione di fine mandato, fine mandato, che hanno l'obiettivo di prendere atto di una situazione di emergenza che ricade anche sulla vita delle amministrazioni locali, che sono veramente il polmone più vicino alla vita dei cittadini. Oggi il nostro dovere è rendere le amministrazioni comunali - e comunque le istituzioni - più vicine ai cittadini, rendere la loro vita più semplice per consentir loro di avere un rapporto con i cittadini più improntato alla soluzione dei problemi, alla vicinanza

È inutile rimanere abbarbicati in una rigidità eccessiva su questioni meramente tecniche, come la relazione di fine mandato o altri adempimenti, e sottrarre tempo alle amministrazioni locali, che invece devono essere il primo sportello per i bisogni dei cittadini. Tanti amministratori che ora sono senatori o che lo sono stati sanno bene

da questo provvedimento dovranno prendere spunto tutte quelle iniziative che devono consentire al Paese di tornare alla normalità. Questo è l'obiettivo che, come classe politica, dobbiamo avere di fronte a noi: nella maniera più rapida possibile questi che sono dei provvedimenti tampone, che cercano di rendere normale ciò che non lo è più; nello stesso tempo, però, come Parlamento dobbiamo dare la spinta e un incentivo forte all'attività del Governo per mettere in campo altri campo altri provvedimenti importanti che devono sostenere la vita economica del nostro Paese. In questi giorni in Senato è in corso l'esame del decreto-legge sostegni, un testo importante che non risolve da solo il problema di tutta quella parte di popolazione che

risposte, che devono essere caratterizzate da un sostegno economico ancora più rilevante di quello che già c'è, e soprattutto dare una prospettiva ordinaria di riapertura a questo Paese. Non si deve creare il partito di chi vuole aprire contro quello di chi vuole chiudere, ma tracciare una strada caratterizzata da programmazione, per vedere quale può essere la via d'uscita, senza creare in questo senso contrapposizioni che non servono a nessuno, che possono alimentare i *talk show,* e non danno risposta a chi fa impresa, a chi deve pagare le bollette e i canoni individuare una strada ben chiara, perché oggi i cittadini vogliono sapere (chi fa impresa, chi ha un negozio, chi ha un ristorante) quando si potranno riaprire le attività, sapendo bene che le condizioni sono dettate dal quadro

provvedimenti che hanno una natura meramente tecnica e - in questo caso - per consentire di svolgere le elezioni tra settembre e ottobre in una condizione di maggiore tranquillità e sicurezza sanitaria; nello stesso tempo, licenziati questi provvedimenti, occorre dare la spinta per il rilancio del nostro Paese, programmare riaperture

per Fratelli d'Italia il voto è il sale della democrazia e in questo momento, particolarmente difficile e sofferto è - a nostro giudizio - anche un elemento ricostituente. Per questo motivo non riteniamo votabile il provvedimento al nostro esame e continuiamo a non capire per quale motivo in tutte le realtà europee si vada al voto mentre In Italia c'è bisogno di spostare la data delle elezioni amministrative. Ci sorge il legittimo sospetto

quale in Italia non si possono tenere le elezioni politiche per effetto della pandemia e, quindi, oggi si sarebbe in enorme difficoltà a far votare i Comuni, perché è ovvio che il virus non fa distinzione. In tal modo, però, noi diamo un ulteriore segnale di allontanamento e di delegittimazione delle istituzioni rispetto alle difficoltà dei cittadini.

Esprimiamo però enorme preoccupazione per come anche il nuovo Governo sta affrontando l'emergenza pandemica in Italia: vaccinazioni a rilento; mancanza di risposte concrete a quelle categorie che stanno pagando più degli altri la difficoltà della crisi, diventata anche economica e sociale. Noi riteniamo gli enti locali, i Comuni e le Province, istituzioni fondamentali nella costruzione del nostro ordinamento statale e voglio esprimere agli amministratori locali tutta la vicinanza e il rispetto del nostro partito nei loro confronti. Sappiamo infatti - e ne siamo consapevoli per essere stati anche noi nella precedente stagione politica amministratori locali - cosa significa stare sui territori ed essere la prima interfaccia dei cittadini, essere investiti di tutte le questioni che in maniera immediata vengono poste a coloro che sono amministratori di prossimità.

abbia ignorato delle questioni che in maniera immediata investono gli enti locali. Abbiamo cercato con una serie di emendamenti di portare il nostro contributo per migliorare

molto discutibili. Ci fa piacere naturalmente che l'attività della Commissione, che voglio ringraziare - e mi riferisco in particolare al mio collega di Gruppo, senatore Totaro - sia riuscita

Sull'emendamento 3.0.11 abbiamo chiesto il voto, perché riteniamo che i sindaci rappresentino l'emblema di quegli amministratori che sono stati caricati di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che hanno già, in tempi ordinari, come autorità sanitaria sul territorio. È incredibile che, rimettendosi a questioni di mero carattere ragionieristico, che rappresentano la morte della politica, non si stia vicino a quegli amministratori che ogni giorno si sbracciano per fare in modo di preservare la propria comunità ed essere vicini ai cittadini più in difficoltà. Tutti gli emendamenti che sono stati proposti, anche dall'ampia maggioranza, confermano che quello in esame era un provvedimento molto carente. Voglio ricordare che i Comuni avevano come problema immediato l'approvazione dei bilanci di previsione e quel e quel problema - noi l'avevamo intravisto, tanto è vero che avevamo proposto un emendamento in proposito - è stato risolto in parte soltanto con un emendamento

In ogni occasione come questa torna nel dibattito la retorica - che tale resta - su tutto quello che si dovrebbe fare e non si fa per per gli enti locali. È evidente che il problema degli enti locali, che occorre affrontare, non è lo spostamento delle elezioni.

I veri problemi, però, non vengono affrontati. Ci sono Comuni che hanno difficoltà finanziarie enormi e cosa si fa? Avevamo proposto un emendamento per sospendere i mutui, per quello che riguarda la quota capitale, con la Cassa depositi e prestiti, che è ciò che incombe maggiormente sui Comuni. Spero dunque che il Governo voglia mettere mano anche a questo aspetto, perché ci deve essere consapevolezza che, soprattutto per dare servizi alle persone, gli enti locali devono avere risorse,

Per quanto riguarda l'aspetto elettorale, bisogna rendersi conto del fatto che ci sono Province il cui mandato è scaduto nell'autunno scorso. Con le nuove norme si arriverà a sessanta giorni dopo le votazioni per le amministrazioni comunali. Aggiungo che non si tratta di una tornata di amministrative come le altre, andranno al voto oltre 1.000 Comuni italiani e, soprattutto, tra essi ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e tante realtà superiori ai 15.000 abitanti.

a cittadini che pagano le tasse esattamente come i cittadini che risiedono nei grandi centri urbani. È stato un gravissimo errore abolire fintamente le Province. La riforma Delrio è stata un fallimento totale perché quel livello istituzionale, il livello di governo in area vasta, è rimasto fantasma. È lì ed è come la nebbia di Totò a Milano: c'è, ma non si vede. Eppure, gestisce servizi fondamentali come l'edilizia scolastica, migliaia di chilometri di strade provinciale che non ricevono interventi di

Credo che sia questa la priorità da affrontare e per questi motivi annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia al provvedimento.

Presidente, in primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento non scontato - come hanno fatto altri - al relatore per il lavoro che è stato fatto in Commissione, così come al Sottosegretario, al Governo tutto e al Presidente della nostra Commissione. Vorrei anche sottolineare che il clima che ha accompagnato nei fatti il decreto-legge in esame è stato davvero estremamente positivo, a basso tasso di intensità polemiche - e questo credo faccia bene a tutti restando sempre su un livello di confronto chiaro, aperto, a cui hanno contribuito tutti: Governo, maggioranza e opposizione. Questo fatto, su una materia così importante e centrale come quella elettorale, è sicuramente una buona notizia, soprattutto se ricordiamo che l'anno scorso andò molto diversamente con il decreto-legge sul rinvio delle elezioni nel giugno 2020. Eravamo convintissimi già allora - lo crediamo ancora di più oggi - che, soprattutto in una fase difficile come questa, il tema elettorale, a prescindere che si parli di *referendum*, Regioni, Comuni più o meno importanti, richiede un dialogo tra Governo e Parlamento; e richiede anche la capacità della maggioranza - anche dell'attuale maggioranza - di coinvolgere l'opposizione, così come, d'altra parte, la disponibilità della minoranza di stare ai fatti e alla realtà, al netto delle battaglie parlamentari che sono sempre legittime in democrazia. Non credo che in quest'anno d'emergenza su questa materia si sia mai adottato un provvedimento contro le opposizioni per opportunità di parte, come di nuovo ho sentito dire anche stamattina da qualcuno il decreto-legge in esame. Credo anzi che lo spirito con cui discusso, e spesso anche migliorato in Parlamento, i provvedimenti che venivano dal Governo sia sempre stato ispirato alla correttezza nonché alla limpidezza. Del resto, i fatti lo hanno dimostrato. ci apprestiamo a convertire oggi si inserisce pienamente in questo quadro: c'è stata discussione in Commissione, c'è stato un dibattito nella sede parlamentare e credo che il confronto alla fine abbia portato a miglioramenti significativi rispetto al testo iniziale, ascoltando soprattutto Comuni, Province, territorio, enti locali. Nel merito, intanto, anche a beneficio di chi ci ascolta, credo sia necessario ricordare e avere presente che noi siamo ancora, purtroppo, in piena emergenza sanitaria. Non possiamo fingere di essere usciti da un periodo straordinario ed eccezionale della storia del Paese e del mondo intero; né possiamo nascondere di venire da un anno e più che ha suscitato preoccupazioni enormi, giustamente, tra i cittadini, che ha provocato lutti in numeri che restano ancora drammaticamente alti, nonostante non siano forse più quelli della fase peggiore, che ha provocato limitazioni, sacrifici duri, direi a dir poco estenuanti per la vita delle persone. Proprio per questo, nonostante la campagna vaccinale sia avviata - e anzi, si possa pensare che già dai prossimi giorni ci sarà una consistente accelerazione nella somministrazione dei vaccini - non possiamo in questo momento abbassare l'attenzione sui rischi che - ad esempio - un turno elettorale si porterebbe dietro. Non potevamo farlo l'anno scorso, quando il turno elettorale - allora comprendeva anche un *referendum* - fu rinviato a settembre, con molte polemiche, anche in Parlamento. E abbiamo visto che quel rinvio non ha portato alcuna minaccia al corretto funzionamento della democrazia e all'espressione della volontà popolare. Non possiamo prescindere da un principio di cautela neanche quest'anno, proprio perché veniamo dall'esperienza delle elezioni del 2020 che, pur svoltesi in modi differenti, hanno garantito il diritto di tutte le forze politiche e di tutti i candidati, oltre che dei cittadini elettori. Per questo, adottando un atteggiamento di prudenza giusto, questo decreto-legge aggiunge un pezzo importante alla costruzione di una nuova normalità che sta ispirando tutti i provvedimenti e tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo nelle ultime settimane e nei mesi passati. Il decreto-legge che oggi convertiamo quindi visto in siffatto percorso, e per questo noi del Partito Democratico lo riteniamo assolutamente rilevante e degno di nota, anche perché in autunno dovranno recarsi al voto poco meno di 1.300 Comuni, tra cui molti tra i maggiori capoluoghi, e un'importante Regione del Mezzogiorno come la Calabria, oltre al voto per le suppletive. Quello oggi all'esame è un decreto-legge che cerca di blindare, nella maniera più corretta possibile, la necessità di garantire lo svolgimento democratico di consultazioni elettorali che erano previste per la primavera e di farlo non solo nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ma anche in un quadro della diffusione dei rischi che si può immaginare ci auguriamo - sia migliorato tra settembre e ottobre. Ecco perché la scelta di tornare a votare su due giorni, soprattutto a tutela dei più anziani, ovviamente. Ecco perché la scelta di farlo in una finestra temporale tra il 15 settembre e il 15 ottobre, che dovrebbe consentire a tutte le forze politiche di presentare liste in tempi ragionevoli e di fare campagna elettorale in modo adeguato. Non si tratta di altro se non di quella linea di prudenza, di principio e precauzione che giustamente questo Governo sta seguendo, peraltro in assoluta continuità con l'impostazione del Governo precedente, che ha dato buoni risultati di efficacia già nel precedente turno elettorale del settembre 2020. Inoltre, con un consenso ampio da parte di tutte le forze politiche in Commissione affari costituzionali, sono state anche rinviate le elezioni per il rinnovo degli organi delle Città metropolitane, per i Presidenti di Provincia e per i Consigli provinciali che scadono nei primi nove mesi del 2021, anziché soltanto nel primo semestre, come era già previsto. In questo modo il rinvio viene correttamente esteso anche a quelle Provincie i cui organi scadono nel mese di luglio. Le elezioni non sono soltanto il giorno in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi con la scheda elettorale, ma sono anche un percorso articolato e complesso. In questo percorso complesso c'è una fase che presenta ovviamente rischi legati agli assembramenti o comunque a possibili

come è stato già nel 2020, basterà soltanto un terzo delle firme attualmente previste per poter presentare le liste. Come Partito Democratico abbiamo condiviso l'esigenza per i Comuni fino a 15.000 abitanti di affrontare il tema dello spopolamento diffuso, che tutti ben conosciamo, e quello del voto degli aventi diritto iscritti all'AIRE. Secondo noi, è giusto affrontare questi punti, soprattutto in questa fase, in cui gli spostamenti tra distanze maggiori o minori sono resi molto difficili. La soluzione è nota: per tutto il 2021, in caso di lista unica, potranno essere eletti tutti i componenti della lista se il numero di votanti sarà del 40 per cento degli iscritti alle liste.

nella nostra Commissione. Abbiamo poi affrontato - come era doveroso - il tema di tutti gli oneri amministrativi per la presentazione delle liste, affidandone per ora la definizione a un ordine del giorno condiviso. Credo altresì che sia importante ricordare l'altro ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutte le forze politiche per la proroga dei permessi ai sindaci, per cui il Governo si è impegnato a inserire una specifica norma nel prossimo decreto-legge, che io credo dovrebbe davvero servire a risolvere alcune difficoltà o dubbi interpretativi pure emersi in questi mesi. Ricordo che stiamo parlando di sindaci che in molte occasioni stanno facendo sforzi davvero straordinari - e a loro vanno il nostro sostegno e la nostra vicinanza, anche personali in comunità di ridotte dimensioni, alle quali lo Stato ha il dovere di far sentire concretamente la propria vicinanza e il proprio supporto, sempre. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, perché è equo ed equilibrato e aggiunge un mattone fondamentale per la costruzione di quella normalità, seppure ancora drammaticamente parziale, necessaria per un appuntamento importante per tante, tantissime comunità del nostro territorio.

con convinzione siamo qui oggi a votare per convertire in legge il decreto-legge n. 25 del 5 marzo del 2021 per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, prevedendo una finestra elettorale tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Consentitemi però di esprimere innanzitutto la mia solidarietà e quella delle senatrici e dei senatori del Gruppo Misto al ministro della salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini *(Applausi)*, vittime entrambi di minacce e intimidazioni, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, con modalità diverse. Si tratta di un clima di tensione pericoloso: basti pensare alla bomba *molotov* all'Istituto superiore di sanità. Ministro Speranza, presidente Bonaccini, noi stiamo con voi. Eccoci al provvedimento che stiamo per licenziare in prima lettura, che ricalca un'iniziativa analoga presa l'anno scorso e che ritengo doveroso, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di varianti del virus che in alcuni casi, come la variante inglese, presentano un carattere anche di maggiore contagiosità. Il decreto-legge prevede - lo abbiamo già sentito - che le consultazioni si svolgano in due giornate. Devo dire che il relatore, il collega Pagano, ha già illustrato ampiamente in Aula i contenuti del provvedimento, e posso dirvi che abbiamo lavorato bene come maggioranza in 1a Commissione. Colleghe e colleghi - come sapete - si sarebbe dovuto votare a maggio per le regionali in Calabria, per i Consigli comunali di città importanti e popolose come Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna (solo per citarne alcune). Tutti avremmo voluto che si fosse votato secondo la scadenza naturale, ma non è stato possibile perché siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Nessuno in quest'Aula può contestare l'evidenza: abbiamo difficoltà nel piano vaccinale; le terapie intensive e i reparti ospedalieri sono occupati oltre la soglia critica; non sappiamo ancora se abbiamo raggiunto il picco dei contagi. Certo, ci sono dei timidi segnali che ci fanno ben sperare, ma il Paese è ancora diviso tra zone rosse e zone arancioni. Abbiamo 550.000 persone attualmente contagiate e ogni giorno contiamo, purtroppo, centinaia di vittime (296 l'altro ieri, 421 ieri). Siamo quasi a 112.000 persone morte in poco più di un anno. Ecco perché ci sembra così irreale il dibattito di questi giorni, alimentato da dichiarazioni di esponenti politici che si oppongono alle misure di contenimento della pandemia da parte del Governo, pur facendo parte della stessa maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Ci sono Regioni che spingono per riaprire e il *leader* della Lega che dice no all'ideologia del rosso. Ma davvero, senatore Salvini, lei è convinto che ci siano fautori dell'ideologia della zona rossa? E a che scopo? Non è il momento di dividerci tra rigoristi e aperturisti. Il presidente Draghi, il ministro Speranza, l'intero Governo e quindi anche i Ministri della Lega dicono una cosa semplice e ovvia: se caleranno i contagi, ridurremo le costrizioni. Sovraesporre un Ministro è sbagliato; personalizzare lo scontro è doppiamente sbagliato; cavalcare la rabbia è sbagliato; lasciare solo chi è in trincea è sbagliato. Non può essere la convenienza a far decidere le eventuali riaperture: riapriremo quando ce lo dirà la scienza e quando ce lo diranno i dati medici. Sappiamo bene che il Paese si sta impoverendo e siamo tutti ben consapevoli che migliaia e migliaia di persone soffrono la crisi economica: quasi un milione di posti di lavoro persi - soprattutto per le donne - a causa delle conseguenze economiche della pandemia e delle restrizioni per contenere i contagi, secondo i nuovi dati diffusi ieri dall'Istat; ieri dall'Istat; tassi di disoccupazione giovanili al 31,6 per cento, nonostante il blocco dei licenziamenti. Avremmo dovuto fare di più, certo. Serviranno altre risorse per fronteggiare zone rosse e zone arancioni. Dobbiamo ancora stringere la cinghia nelle prossime settimane. Rivedremo la luce solo quando avremo sconfitto la pandemia. E, quando l'avremo sconfitta, dovremo rimettere al centro il lavoro (quello del nuovo modello di sviluppo), *recovery plan*, transizione ecologica e digitale. Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli suddivisi in sette commi. L'articolo 1 dispone il differimento per l'anno 2021 delle tornate elettorali, spostandole tra il 15 settembre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. In Commissione affari costituzionali è stato svolto un proficuo lavoro migliorativo del provvedimento. Mi limito a segnalare solo un elemento su cui non è stato possibile intervenire: si tratta del tema dei permessi lavorativi dei sindaci, che coinvolge in particolare i sindaci dei Comuni di piccola dimensione. Infatti, nei Comuni di minore dimensione demografica la gran parte dei sindaci sono lavoratori dipendenti che si sono trovati oggi ad affrontare una situazione di emergenza inaudita. Per le stesse motivazioni per le quali era stata prevista la possibilità la possibilità di usufruire fino a ventiquattro ore di permessi ulteriori rispetto alle quarantotto ore previste in regime ordinario dal testo unico sugli enti locali, sarebbe opportuno ripristinare la possibilità di usufruire delle settantadue ore di permesso fino alla fine della cessazione dello stato di emergenza, come da proroghe intervenute o che interverranno. Ci permettiamo di segnalare, quindi, al Governo questo elemento da considerare nei prossimi provvedimenti. Presidente, Governo, colleghe e colleghi, mi accingo a concludere l'intervento. C'è un ultimo punto che vorrei toccare. Mi rivolgo ancora una volta al Governo. Abbiamo bisogno di abbattere il muro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo essere in prima linea nella mobilitazione per chiedere l'universalità dei brevetti sui vaccini e la sospensione della proprietà intellettuale per poter produrre dappertutto e nel numero di dosi necessarie. Vorrei citare il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano: «Più il virus si replica e più genera varianti. Dobbiamo fermare la corsa del virus. Dobbiamo impedire che circoli, qui e altrove». Il virus circola nei Paesi ricchi e nei Paesi poveri e ciò vuol dire che senza vaccini nei Paesi poveri saremo sommersi dalle varianti. La salute è un bene comune; la salute è un diritto, non un privilegio. Presidente, per questi motivi e per l'urgenza e utilità di questo decreto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,

posto all'attenzione per primo in questa discussione dal senatore Astore e poi ripreso anche dalla collega Pirovano. È arrivato il momento - è questo il momento opportuno - di ripensare a quella famosa riforma Delrio, che abbiamo sempre contestato perché crediamo che la democrazia non abbia un prezzo, perché crediamo che la rappresentanza non debba essere sacrificata sull'altare dei tagli economici, perché crediamo che il cittadino ha bisogno di avere un rappresentante di prossimità oggi più che ieri, visto che c'è stato un irrazionale e irragionevole taglio dei parlamentari che fa diventare i consiglieri comunali, i sindaci e i consiglieri provinciali i primi interlocutori dei cittadini. Il Parlamento si allontana dai cittadini e allora diamo forza e dignità alle istituzioni intermedie. Ben venga, quindi, il convincimento degli amici del Partito Democratico che hanno capito meglio - *melius* *re perpensa* - che quella riforma forse poteva avere un senso in prospettiva della riforma costituzionale. I cittadini, però, hanno bocciato quella riforma costituzionale e noi abbiamo non il diritto, ma il dovere di rimettere le cose a posto. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a parlarne da subito e a mettere le cose a posto. Un'altra questione, che pure è stata trattata e che ci vede assolutamente d'accordo, è prevedere il terzo mandato per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Non bisogna essere dei politici di professione per capire quanto sia difficile oggi trovare persone disponibili a sacrificare tempo, famiglia e lavoro nell'interesse del territorio. *(Applausi)*. Pertanto, quando questo è possibile e quando questa persona perché dobbiamo cancellare esperienze, intelligenze e disponibilità, visto che, comunque, non sono delle chiamate dirette, ma c'è sempre un vaglio da parte dei cittadini e degli elettori? Ben venga, allora, anche la discussione, senza riserve e senza pregiudizi, sul terzo mandato per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Voglio dire qualcosa sull'intervento fatto dal collega Ruotolo a proposito delle riaperture e delle posizioni che, anche all'interno di questo Governo, vengono espresse in piena libertà e con assunzione di responsabilità. Chi vi parla non è sicuramente un negazionista: e vorrei vedere chi può negare una pandemia così virulenta, che ha prodotto più di 110.000 vittime! evidente che il Comitato tecnico scientifico, che è fatto di scienziati, darà il disco verde quando la pandemia sarà completamente debellata. La politica ha un'altra responsabilità. La politica ha la responsabilità di decidere, di tenere conto degli scienziati e delle loro valutazioni, ma di decidere. decidere. Non è possibile che nel nostro Paese, per evitare di morire di pandemia si debbano creare le condizioni per morire di fame. *(Applausi)*. Credo che dopo un anno, dopo 110.000 morti, ci sia la possibilità di trovare dei protocolli che possano consentire, consentire, con raziocinio e con intelligenza, di riavviare le attività produttive. Perché nei ristoranti non si può cenare e invece si può cenare negli alberghi? Perché questa discriminazione? I problemi dell'assembramento si risolvono mettendo mano alla movida. Sono i giovani - e se ne capisce il motivo - i più recalcitranti al rispetto delle regole.

Non possiamo aspettare di debellare completamente la pandemia per riaprire, perché, dopo la pandemia, avremo una gravissima crisi economica, che, probabilmente, non saremo in grado di fronteggiare. Quelli che chiamiamo ristori, sostegni e supplenze sono, infatti, gocce nel mare, che non fanno altro che mortificare coloro che, da un anno, hanno chiuso i battenti.

Voteremo quindi questo decreto-legge, che nasce per le stesse motivazioni per cui è nato questo Governo. L'attuale Governo è nato per l'inopportunità di andare al voto in un momento nel quale, probabilmente, il voto avrebbe potuto creare un elemento di aggravamento della pandemia. Giustamente, come conseguenza, anche le elezioni amministrative sono state rinviate, in un momento nel quale ci auguriamo che, partendo come si deve la campagna di vaccinazione, con una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e rigidi protocolli sanitari, che si possono senz'altro anche il diritto costituzionale di esercitare il proprio voto, sia pure in amministrazioni e in organismi intermedi, possa essere esercitato. Qualche modifica è stata accettata in Commissione. Noi abbiamo cercato di portare un contributo, visto che ci trovavamo in un momento delicato, per riflettere su alcune storture

dell'irragionevolezza (molte volte) delle norme legislative. Viene posta una sanzione a carico del partito che non ha provveduto, nei quindici giorni precedenti al voto, a pubblicare sul proprio sito il certificato penale dei candidati. le liste vengono presentate trenta giorni prima ed è irrazionale prevedere una sanzione quando ormai il termine per la presentazione delle liste è evaporato: ed è irrazionale soprattutto quando il partito dimostra documentalmente di aver richiesto il certificato il certificato penale al cittadino. Ci è stato detto dal Sottosegretario che questa non era la sede per affrontare il tema e che forse la normativa era troppo giovane per essere sottoposta a una rivisitazione

anche dire agli amici dei 5 Stelle, che hanno fatto di questa norma un cavallo di battaglia, che nessuno vuole sottrarre i partiti alla responsabilità della trasparenza nelle candidature e nella designazione dei loro rappresentanti; ma facciamo una normativa razionale,

nel momento in cui si devono presentare le liste, con i tempi ristretti, gli imprevisti, gli inconvenienti, le sostituzioni, le rinunce e le nuove candidature. È impossibile tenere conto di tutto questo in maniera ragionevole e razionale.

all'interno di città che sono state gravemente colpite dalla pandemia e che quindi più delle altre hanno subito le difficoltà e l'emergenza. Ma, come diceva qualcuno oggi in Commissione, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole, con la consapevolezza che questo è soltanto il primo passo per cercare di porre rimedio a tante storture e a tante normative che hanno dimostrato...

il decreto-legge che andiamo oggi a convertire tocca un tema estremamente delicato: il rinvio delle elezioni, ossia di ciò che sta alla base di ogni sistema democratico. Il Governo interviene per decreto per posticipare non solo i rinnovi delle amministrazioni locali, ma anche di tutti i seggi vacanti nel Parlamento. Il potere Esecutivo quindi interferisce di fatto su quello legislativo e ciò è sicuramente l'elemento costituzionalmente più rilevante del decreto-legge n. 25. Il passaggio di ratifica parlamentare non è quindi un semplice atto dovuto, ma è il momento e il luogo in cui è indispensabile compiere un'attenta valutazione circa la portata degli elementi positivi e negativi del quadro di insieme in cui ci troviamo. Lo stato della pandemia non ha impedito ad altre nazioni di procedere diversamente. Importanti elezioni si sono tenute nelle scorse settimane e altre ne verranno nel corso della primavera; quindi nel bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla democrazia ha prevalso la scelta di non comprimere quest'ultimo. Il nostro Paese invece, che - lo ricordo - è stato il primo a scontrarsi con gli effetti del Covid, sembra destinato a essere tra gli ultimi a uscirne, a causa di un piano vaccinale male impostato e fatto partire lentamente e in colpevole ritardo, in cui si è data priorità alle coreografie delle primule e non all'approvvigionamento di vaccini e alla disponibilità di personale sanitario. Per fortuna, con la destituzione del commissario Arcuri e l'arrivo del generale Figliuolo, il *trend* è cambiato e si procede a recuperare il tempo perduto confidando di raggiungere l'obiettivo nel corso dell'estate. Diventa quindi concepibile un rinvio delle previste elezioni, non di un anno, ma di quindici settimane, per permettere al Paese di affrontare la campagna elettorale con maggiore serenità e senza troppi vincoli e limitazioni. Queste sono le premesse che portano il nostro Gruppo a dichiarare il voto favorevole e ad accettare questo slittamento dei termini per l'esercizio di un diritto fondamentale come quello del voto. Sarebbe difficilmente attuabile un rinvio ulteriore, perché città importanti come Roma, Milano, Torino e Napoli necessitano di un rinnovo e di un rilancio della vita amministrativa e l'accanimento terapeutico nel tenere in vita le Giunte Raggi, Sala, Appendino e De Magistris sarebbe l'ulteriore punizione per milioni di nostri concittadini. Purtroppo dovremo trascinarci anche la ridicola e stucchevole *soap opera* con la quale la sinistra crede di tenere col fiato sospeso il Paese. Dovremo attendere l'autunno per sapere chi sarà il loro candidato paracadutato nel collegio di Siena alla Camera: Sarà Conte? Sarà Letta? Una manfrina infinita, che prende in giro gli elettori senesi, che invece meriterebbero rispetto e di essere rappresentati da un parlamentare che conosca il territorio e che sia ad esso legato. Il passaggio parlamentare di questo decreto è stata però l'occasione per inserire alcuni correttivi indispensabili per le elezioni comunali nei piccoli Comuni. Lo affermo con soddisfazione, perché la Lega è da sempre al fianco di queste realtà ed è attenta, come nessun altro, alle loro necessità ed esigenze, anche grazie al fatto che molti senatori del Gruppo della Lega sono prima di tutto amministratori locali. Anche grazie al costante confronto e al dialogo con l'Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia e con la sua instancabile presidente, Franca Biglio, nonché con il responsabile del Dipartimento piccoli Comuni ANCI, Massimo Castelli, siamo riusciti a proporre soluzioni condivise da tutti a problemi presenti da tempo. I piccoli Comuni non sono una nicchia: sono ben 5.500 su 7.900; ben il 70 per cento dei sindaci è sindaco di un piccolo Comune e solo nella Regione Lombardia e in Piemonte se ne contano più di 2.000. Nei piccoli Comuni abita un connazionale ogni sei e, con più di 10 milioni di abitanti, si tratta di fatto della Regione più grande d'Italia: una popolazione grande come quella della Grecia, della Svezia o del Portogallo. È amministrato dai piccoli Comuni il 54 per cento del territorio nazionale e quasi la totalità delle nostre bellezze naturali è nelle mani di sindaci che hanno sempre meno strumenti e sono sempre meno motivati nel proseguire il loro impegno che, di fatto, è unicamente di volontariato sociale. Molti piccoli Comuni rischiano ora di trovarsi senza amministratori per la difficoltà, accentuata dal Covid-19, di raggiungere il *quorum* di validità richiesto quando a presentarsi alle elezioni è una sola lista.

Mentre per le elezioni nazionali e i *referendum* è previsto il voto per corrispondenza su circoscrizioni indipendenti, per le amministrative l'unico modo per votare è in presenza, con un viaggio magari intercontinentale: in ogni caso, l'elettore concorre a determinare il *quorum*. Vi porto a conoscenza di uno degli infiniti esempi che potrei fare, quello di un Comune delle Prealpi vicentine, Posina. Alle elezioni dello scorso settembre risultavano iscritti 1.149 elettori per le comunali e 459 per il *referendum* nazionale. La differenza di 700 votanti, più della metà, è data appunto da elettori AIRE. Ebbene, al voto si sono presentati in 357, che hanno ritirato entrambe le schede. C'è stato il 78 per cento di affluenza per il *referendum*, ma il 31 per le comunali. Se non fossero state presentate più liste, quelle elezioni sarebbero state annullate e il Comune sarebbe stato commissariato. In casi come questi è matematicamente impossibile raggiungere il *quorum* con i soli elettori realmente residenti. Abbiamo così proposto di abbassare la soglia al 40 per cento e, soprattutto, di escludere gli elettori AIRE dal calcolo del *quorum* di validità. Con il voto favorevole al nostro emendamento di poco fa abbiamo dato respiro e futuro a tante piccole comunità. La norma avrà effetto straordinario per le elezioni 2021, ma confidiamo di metterla a regime a breve con apposito disegno di legge già in fase avanzata di esame. Con lo stesso disegno di legge c'è la volontà di porre fine al fenomeno delle liste fantasma, ossia quelle liste di candidati ampiamente estranei alla comunità e che, unicamente per trarre vantaggi personali sotto forma di permessi retribuiti e periodi di aspettativa, mettono in seria difficoltà anche economica i Comuni con meno di 1.000 abitanti, sfruttando la possibilità di non dover raccogliere sottoscrizioni di elettori al momento del deposito delle liste.

irrisolta la duplice problematica del terzo mandato consecutivo dei sindaci. Questa possibilità è concessa ora solo ai micro Comuni con meno di 3.000 abitanti ed è vietata a tutti gli altri, chiediamo che venga estesa a tutti i Comuni fino a 15.000 abitanti. Chiediamo altresì che venga corretta la norma che consente un massimo di tre mandati totali ai sindaci dei micro Comuni. Quest'anomalia normativa porta infatti a una forte diseguaglianza, in quanto il sindaco di una metropoli può essere eletto per quattro mandati, alternati da un turno di pausa dopo due in carica, mentre il sindaco di un Comune di 200 persone è per sempre ineleggibile dopo un totale di tre turni. Il rischio concreto è di non trovare più persone capaci e disponibili che scelgano di mettersi al servizio della collettività, disperdendo così l'esperienza amministrativa maturata. Ciò è tanto più vero in una fase storica come quella dell'emergenza Covid, che ha messo a dura prova i sindaci, i quali si sono ritrovati spesso ad essere l'unico punto di riferimento della loro comunità.

Nel ringraziare chi ha operato per il buon esito dell'esame in Commissione (il presidente Parrini, il relatore Pagano e il sottosegretario Scalfarotto, a dimostrazione della possibilità

Sin dalla nascita della Repubblica italiana questo tema è uno di quelli rimasti uguali a se stessi nel tempo. Infatti, le elezioni si svolgono esattamente nello stesso modo di come si facevano nel 1948 e - anzi - di come si tenevano all'inizio del secolo e nell'Ottocento. modo, tutte le procedure di presentazione delle liste sono rimaste inalterate e - lasciatemi dire - estremamente e inutilmente farraginose. Se, da una parte, le elezioni sono il pilastro fondamentale della nostra democrazia, dall'altra sono l'istituto che fino a oggi ancora non ha saputo cogliere gli elementi positivi offerti dalla digitalizzazione per poter snellire, sburocratizzare e rendere più sicuri i propri processi. Conosco bene tutti questi temi perché da anni mi occupo in prima persona di organizzare i rappresentanti di lista per il MoVimento 5 Stelle nella Provincia di Modena, supportando anche il lavoro nelle altre Province dell'Emilia-Romagna. Chi, come me, fa questa attività (che potrei definire di supporto alla democrazia) sa bene come spesso sia la burocrazia stessa a fungere da argine alla trasparenza. in discussione oggi tocca solo marginalmente questa materia, spostando in avanti nel tempo la tornata elettorale amministrativa prevista per questa primavera. un atto evidentemente necessario, visto che la campagna vaccinale è in pieno svolgimento e si è ancora alle prese con la terza ondata della pandemia. Tra l'altro, andranno al voto città come Roma, Bologna, Milano, Napoli e Torino, solo per citare le più popolose. Per questo motivo è importante garantire una campagna elettorale che sarebbe stata impossibile assicurare il prossimo mese. Credo sia però necessario andare oltre il semplice differimento delle elezioni e ragionare su alcune modifiche strutturali che possono essere utili all'Italia in qualsiasi momento storico

l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato stesso. In quest'ultimo anno, abbiamo definitivamente sdoganato la necessità di inviare documenti, accedere a sussidi e a procedure amministrative tramite piattaforme digitali. L'esempio della crescita esponenziale delle attivazioni dello Spid da parte degli italiani ne è la testimonianza più tangibile. Di fronte a questo cambio di paradigma, com'è possibile che un atto semplicissimo come la presentazione dei nominativi dei rappresentanti di lista debba ancora avvenire in forma cartacea, magari facendo spostare le persone decine di chilometri per farla? Il sistema Spid è utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e comunali. Credo sia ora che si introducano sistemi informatizzati anche per espletare la presentazione di documenti per motivi elettorali. Il mio emendamento adesso è limitato solo a questa tornata elettorale autunnale e dà la possibilità, entro il mercoledì antecedente alle elezioni, di inviare le nomine dei rappresentanti lista con una PEC. In futuro, spero si possa allargare la fascia temporale arrivando fino al venerdì antecedente il voto e che si renda strutturale l'utilizzo della PEC per questo tipo di comunicazioni. In questo senso ho depositato un disegno di legge, atto Senato 2129, assegnato alla 1a Commissione, che va proprio in questa direzione, attorno al quale spero convergano i pareri positivi da parte di tutte le forze politiche. Ringrazio il presidente Parrini per la sottoscrizione ed il sostegno. Devo rilevare come tutte le discussioni intorno alle elezioni negli ultimi tempi si sia focalizzata a mio modesto avviso su obiettivi sbagliati o comunque fuorvianti. ad esempio, ad una diatriba dialettica intorno alla necessità di allargare il voto ai sedicenni, un tema importante e da approfondire sicuramente, sicuramente, ma credo che lavorare sulle procedure, sulla burocrazia legata alle elezioni sia l'azione necessaria da compiere per stare al passo coi tempi. fa meno notizia parlare di procedimenti di riforma del processo elettorale rispetto ad altro, ma bisogna fare lo sforzo di non farsi distrarre per migliorare definitivamente l'*iter.* Un altro intervento che mi riprometto di portare avanti in questa legislatura è la proposta di chiusura anticipata dei seggi elettorali rispetto al canonico orario delle 23. Chiudere alle ore 22 mi pare più corretto. Chi ha fatto parte dell'ufficio elettorale di sezione è consapevole della quasi inoperosità degli stessi dopo le ore 22. Se guardiamo all'esempio della maggior parte dei nostri *partner* europei, i seggi vengono chiusi molto prima. Di questo beneficerebbero le operazioni di voto, gli scrutatori e la velocità con cui avere i risultati. Lasciatemi aggiungere che sarebbe anche una necessaria cortesia di comunicazione e trasparenza verso l'elettore quella di far uscire i risultati già consolidati entro la mezzanotte. Infine, ma non meno importante, si avrebbe un risparmio per le casse dello Stato, perché al massimo il giorno dopo la chiusura dei seggi si chiuderebbero tutti gli scrutini. in questa legislatura storica abbiamo portato a termine riforme epocali come la riduzione del numero dei parlamentari, che contribuiscono a rendere più snello l'apparato politico italiano. È il momento di fare un passo avanti anche sulle elezioni, che devono diventare finalmente 2.0. La tecnologia è una nostra alleata e non deve essere vista con diffidenza. Questo non è un passo solo per noi stessi, ma per i nostri figli che guardano con sgomento un procedimento elettorale vetusto, interrogandosi sull'utilità di questo spreco di carta e dei relativi aggravi burocratici che ingabbiano le loro intelligenze. Permettetemi, in conclusione, un riferimento al singolare caso delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza che i prossimi 18 e 19 aprile rischiano di doversi svolgere in presenza. Per questo chiedo nuovamente al presidente della mia Regione Bonaccini e all'assessore Mammi di attivarsi immediatamente al fine di rinviare queste elezioni evitando la convocazione di quasi 150.000 persone. Mi avvio alla conclusione auspicando che in prospettiva, quando si potrà tornare al voto in sicurezza, gli aventi diritto vadano ad esercitare il diritto-dovere di votare, perché come diceva David Foster Wallace avete tutto il diritto di stare a casa se volete, ma non prendetevi in giro pensando di non votare. In realtà, non votare è impossibile, si può votare votando oppure votare rimanendo a casa e raddoppiando tacitamente il valore del voto di un irriducibile. Concludo con l'auspicio che in tempi brevi si possa procedere alla digitalizzazione e al taglio dell'inutile burocrazia anche per quanto attiene al farraginoso procedimento elettorale e annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame.

All'articolo 2, comma 1-*bis,* introdotto dall'emendamento 2.4, al primo periodo, si propone di sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti»; al secondo periodo sostituire le parole: «qualora non sia raggiunta tale percentuale» con le seguenti: «qualora non siano raggiunte tali percentuali». Al comma 1-*bis,* introdotto l'emendamento 2.5, si propone di sostituire le parole: «per le prossime competizioni elettorali» con le seguenti: «per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti».

«prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021». *al comma 2, sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* essendo modificato il provvedimento con l'introduzione di emendamenti in Commissione e votati già in Aula, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali», si propone di inserire le seguenti: «, nonché relatore, mi sembra inusuale una così lunga Il problema è che non siamo in grado di capire se si tratta di semplici correzioni formali o di correzioni sostanziali.

Se il relatore insiste, prima di dare per assodato che non si tratti di correzioni sostanziali,

Non basta un'accelerazione unanime.

Signor Presidente, finalmente, in un'Aula deserta, arriva la mozione, presentata il 26 gennaio sottoscritta e fortemente voluta anche dai colleghi di Lega e Forza Italia, per un totale che ha superato un quinto dei membri presenti in Senato, il che avrebbe dovuto darle il diritto alla procedura abbreviata, ovvero la discussione entro trenta giorni. Ciò non è non è stato rispettato il Regolamento del Senato. Soprattutto, ricordo almeno quattro Conferenze dei capigruppo in cui Fratelli d'Italia ha chiesto la calendarizzazione della mozione, ma la respinta. Ecco perché dico che oggi finalmente arriva in Aula. Veniamo al merito, perché ho pochi minuti e spero di convincere anche i riottosi sorprendentemente riottosi - che la suddetta mozione non solo è una proposta fattibile, di buon senso, utile e necessaria, ma aggiungerei che è attesa da chi è fuori di qui. La contestualizzo velocemente. La legge di bilancio del 2020 ha previsto di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, il Piano Italia *cashless*, ovvero un rimborso in denaro per le spese effettuate con tali strumenti. All'interno del piano, la misura più popolare è proprio quella del *cashback*, ovvero del rimborso del 10 per cento su transazioni effettuate con moneta elettronica con un massimale di 150 euro. Per il *cashback*, il Governo ha stanziato

misura non ha ottenuto gli effetti sperati, ma soprattutto il *cashback* non risponde alla finalità dichiarata, ovvero quella di rappresentare uno strumento di lotta all'evasione fiscale: è come minacciare con una pistola ad acqua.

ovvero il *cashback*, secondo la BCE, non terrebbe nella debita considerazione che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che per varie - legittime - ragioni preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Questo lo dice la BCE, non lo diciamo noi. Vengo agli impegni del Governo. La mozione impegna il

Ci si assume la responsabilità se sostenere concretamente le categorie e le attività chiuse per Covid-19, aggiungendo 5 miliardi a quegli insufficienti e mortificanti 11 miliardi dei ristori (briciole, rispetto ai danni); la responsabilità di non aver dato una *roadmap* per la riapertura; ci si assume la responsabilità del fallimento di alcune imprese, costrette ancora a pagare costi fissi come affitti e bollette.

la mozione si assume la responsabilità di rispondere: non vi lamentate, avete la riffa, la lotteria degli scontrini e lo spreco vergognoso del *cashback* (che qualcuno ha deciso di non dare a chi lo merita, a chi soffre, a chi sta per chiudere, a chi fa sacrifici e a chi non ha più pane). Pur condannando le violenze di alcune manifestazioni, non si può non condividere l'esasperazione e non provare solidarietà verso chi è stato chiuso per decreto, non è stato indennizzato e non sa cosa mettere in tavola per i figli ogni giorno. Mettetevi una mano sulla coscienza, quando voterete oggi. finestra"). Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, dei senatori Dell'Olio, Bagnai, Errani, Manca, Conzatti, Damiani, Steger ed altri,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sommessamente ricordare quale sia il periodo storico in cui il Governo ha scelto di implementare una misura superflua e ideologica (ideologica perché naturalmente chi utilizza il contante è sempre e comunque uno sporco evasore) come il *cashback* e di metterci sopra 5 miliardi miliardi di euro. Nell'anno appena trascorso abbiamo visto morire in Italia 300.000 imprese a causa della gestione della pandemia, che è stata sempre e solo di chiusure. La pandemia è stata gestita così dal Governo giallorosso, che era il Governo dei peggiori, ma la gestione è stata replicata, pari, pari, anche dal cosiddetto Governo dei migliori. Ricordo - perché ci ci pare che questo Governo sia un po' distratto - che nel 2020 il sistema produttivo italiano ha avuto un calo di fatturato di 423 miliardi,

ha voluto "rimediare" - il termine, per chi non lo capisse, naturalmente è ironico e credo che non ci sia mai stata ironia più tragica di questa - con un totale di contributi a fondo perduto pari a 11 miliardi Vorrei che queste due cifre, 423 miliardi e 11 miliardi, si scolpissero bene nella testa di tutti (soprattutto le proporzioni). Signori e membri del Governo, prima di alzare il sopracciglio dai nostri scranni privilegiati perché ieri qualche ristoratore e qualche commerciante

sono molto stupita che queste proteste arrivino solo ora, dopo un anno di coma economico del nostro sistema produttivo,

Le persone di ieri - dobbiamo ricordarlo - non sono professionisti della protesta e non appartengono ai centri sociali, ma pensano che non rialzeranno mai più la loro serranda, non sanno cosa dare da mangiare ai loro figli domani e hanno visto polverizzare in un anno il sudore, le lacrime e i sogni di una vita intera. E voi - perché Fratelli d'Italia, è bene sottolinearlo, non ha alcuna responsabilità in questa vostra "follia", e non saprei usare un sostantivo diverso invece di destinare ogni centesimo disponibile ai rimborsi per queste persone, concedete ristori, come un sovrano concede ai sudditi. Destinare 5 miliardi al *cashback*: per noi siete dei marziani. Non sentite vergogna morale dentro di voi? Non capite la vostra miopia sulla visione economica della nostra Nazione?

cancelli subito questa follia modaiola e ideologica del *cashback* e metta 5 miliardi per lenire - certo, parzialmente - le ferite di quell'Italia che lavora (o, forse, sarebbe più giusto dire che lavorava).

le finalità attribuite alla misura del *cashback* sono due: l'aumento della digitalizzazione delle transazioni effettuate nel nostro Paese e la diminuzione dell'evasione fiscale. Possiamo già in parte misurare alcuni effetti legati al primo obiettivo, perché sappiamo quante sono le transazioni effettuate le transazioni effettuate (circa 7,2 milioni) e sappiamo anche che sono quasi 15 milioni gli strumenti elettronici di pagamento attivati per poter beneficiare di questa misura.

a maggior ragione per quanto riguarda una misurazione degli effetti della riduzione dell'evasione fiscale. Non è pensabile che in soli tre mesi si possa stabilire se questa misura abbia avuto un effetto positivo positivo o meno sull'emersione del nero. È inutile che ce lo nascondiamo: sappiamo bene che in molti casi i pagamenti vengono effettuati in una modalità che non permette la tracciabilità e, quindi, con comportamenti poco ortodossi. Credo che, proprio per il breve lasso di tempo che ci separa dall'introduzione di questa misura e dall'avvio della sua operatività, prima in maniera sperimentale e oggi più ordinata e concreta, abbiamo la necessità di prenderci del tempo per meglio meditare sugli effetti legati alle finalità e ai principi che questa misura si è data. però accorgimenti che già oggi possiamo dirci essere necessari, perché la mole di risorse che stiamo impegnando su questo provvedimento la modalità con la quale si sta sviluppando ci fa dire che possono essere già oggi adottati correttivi che si traducono ovviamente in risparmi. I correttivi possono essere rispetto al numero di transazioni semestrali, al tetto del valore delle transazioni stesse e alla possibilità che anche i commercianti e gli esercenti recuperino almeno in parte i maggiori costi derivanti dalle commissioni sulle transazioni elettroniche. I miglioramenti, che si traducono in risparmi, sono certamente possibili e fattibili. C'è anche il tema che riguarda - ahimè - le operazioni che si fanno in questo Paese: cambiano i Governi e chi arriva dopo passa il tempo a smontare le misure fatte dal Governo e dalle maggioranze precedenti. Uno dei grandi temi del nostro Paese è la certezza del diritto

La certezza del diritto è infatti uno dei capisaldi su cui si basano gli investimenti. I commercianti e gli esercenti che hanno dovuto adeguare i propri sistemi elettronici per poter accogliere queste modalità di pagamento a supporto del *cashback* e dell'altra misura, quella della lotteria degli scontrini, hanno fatto investimenti e, se si dice loro che abbiamo scherzato e che quegli investimenti vanno a decadere, credo che non sia neppure rispettoso dell'impegno che

dovrebbe fare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per far sì che le commissioni sugli strumenti di pagamento elettronici e sulle modalità di introduzione

di transazioni, che è già sensibilmente cresciuto, è facile fare un calcolo del maggiore introito che banche e carte di credito hanno conseguito. Credo allora che il Governo possa aprire una trattativa con l'ABI per poter diminuire in maniera significativa le commissioni su questi strumenti.

la questione del cosiddetto *cashback* ha visto la formazione di un nuovo Governo e, soprattutto, la necessità che le forze politiche tengano conto del percorso che questo Governo si è prefisso. Li conosciamo, ce li ripetiamo spesso e magari non finiscono nelle trasmissioni, più o meno urlate, che si vedono la sera, ma sappiamo perfettamente che l'impulso che è stato dato alla questione dei vaccini dovrebbe indurre un po' tutti noi, tutte le forze politiche, a concentrarci sui numeri e sull'andamento della campagna, perché da quello dipenderanno,

ovviamente in un quadro economico che non è quello che andremo ad affrontare. Ritengo quindi che sia un po' complesso pensare di spostare una somma, che, di fatto, è già in gran parte impegnata, da uno scopo a un altro.

che vediamo tutti i giorni, naturalmente, non solo nelle manifestazioni, ma anche sull'andamento complessivo del piano vaccinale. La questione del *cashback* va corretta, su questo non c'è alcun dubbio, alla luce di alcuni dati. Uno, citato prima dal collega che ha preceduto il mio intervento, è relativo alle commissioni bancarie.

La prospettiva di questo *cashback*, al di là della questione più specifica, spesso richiamata, della lotta all'evasione fiscale, dal dicembre 2020 al dicembre 2022, è quella di dare 24 miliardi di consumi aggiuntivi,

lo è sicuramente, ogni giorno, il controllo delle vaccinazioni che sono state fatte e di quanto stanno andando avanti nel Paese le coperture per deboli e anziani, per poi passare alle altre categorie. *(Applausi)*.

anch'io intervengo rispetto al *cashback*, ricordando che la legge di bilancio 2020, che l'aveva previsto, aveva visto la Lega in una posizione contraria, soprattutto rispetto alla demonizzazione dell'utilizzo del contante. Io per prima utilizzo moltissimo per i miei pagamenti la carta di credito

Un giorno una persona un po' disagiata mi ha detto: «cosa vuoi che mi faccia il bancomat, se prendo 600 euro al mese?».

ha bisogno di un correttivo, viste le necessità derivanti dalla pandemia, fermiamoci e facciamo un monitoraggio per vedere quello che è successo a partire dall'8 dicembre, traendone le conclusioni. Ricordo un articolo de «Il Sole 24 Ore» dell'11 dicembre, che evidenziava molte criticità. È uno strumento nuovo e quindi vediamo come ha funzionato,

che non riesce a fare bene i conti e che alla cassa ha il problema di non avere copertura sulla carta di credito; quindi, in mezzo a un grandissimo imbarazzo,

è mia convinzione che questa mozione non si basi su dati di fatto, numeri, statistiche ed evidenze inconfutabili, ma si inquadri nell'ambito di un più generale contrasto politico, del tutto legittimo peraltro, all'operato di questi anni di Governo del presidente Conte e del MoVimento 5 Stelle, tentando di contestare, ridicolizzare e dileggiare qualsiasi cosa fatta, anche quelle meglio riuscite, come quella di cui ci occupiamo oggi.

I proponenti sottolineano che sarebbe necessario dimostrare che le misure siano realmente efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere e che, quindi, dovrebbe sussistere una chiara e inequivocabile prova che il meccanismo di *cashback* consenta di fatto di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale. Vediamo allora quali sono questi numeri,

una minore circolazione del contante, il che consente significativi risparmi legati alla sua gestione, costo che grava sia sugli operatori economici sia sullo Stato. Si pensi agli oneri delle assicurazioni contro furti o rapine o a quelli della sicurezza, dei controlli anticontraffazione e così via. Aumentano poi i consumi, che da anni sono molto bassi, anche a causa della crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008. C'è poi l'emersione di una parte dell'economia sommersa, con conseguente aumento della base imponibile, che potrà portare a una maggiore efficacia del contrasto all'evasione fiscale e a una diminuzione generalizzata delle tasse. Quali sono ad oggi i dati disponibili di cui possiamo parlare? Una parte ci è stata fornita dal sottosegretario Durigon, della Lega, qualche giorno fa, rispondendo a un'interrogazione alla Camera.

per cento dei pagamenti tra 30 centesimi e 5 euro. A marzo i cittadini iscritti al programma erano oltre 8 milioni, 7 milioni dei quali erano utenti attivi, e gli strumenti di pagamento registrati sono passati dai 9,6 milioni di dicembre agli oltre 14 milioni di marzo. Tra questi, gli strumenti di pagamento attivi sono passati da 6,7 milioni a dicembre a 9,7 milioni a febbraio, con un incremento di circa il 20 per cento di mese su mese: sono sempre dati forniti dal sottosegretario Durigon. Tutto ciò, che è un clamoroso successo, è stato ottenuto in pochissime settimane,

in poco meno di un anno, sono passate dai 5,7 milioni del gennaio dell'anno scorso ai 16,4 del gennaio di quest'anno. Secondo un sondaggio della Community cashless society, il 70 per cento degli italiani pensa che il *cashback* abbia spinto ad un uso più frequente

parere contrario sulla mozione e accoglie l'ordine del giorno che impegna l'Esecutivo ad approfondire il monitoraggio del programma *cashback* anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici, in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

colleghe senatrici e colleghi senatori, membri del Governo, parliamo oggi di un argomento che è stato molto dibattuto nell'ultimo periodo.

bancomat e applicazioni di pagamento. Il rimborso è previsto nella misura massima di 300 euro l'anno, ossia fino a 150 euro a semestre, a fronte di almeno 50 pagamenti. Il rimborso massimo per ogni singola transazione è invece di 15 euro. di 15 euro. A differenza della cosiddetta Lotteria degli scontrini, per il *cashback* non è previsto un importo minimo di spesa e chi partecipa al programma, peraltro, può concorrere anche all'assegnazione del super *cashback,* ossia di un premio in denaro, di importo fino a 3.000 euro, che viene concesso ai primi 100.000 cittadini che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamenti elettronici. La misura era stata lanciata in via sperimentale nel dicembre dello scorso anno con il cosiddetto *cashback* natalizio, però è solo dal gennaio 2021 che questo strumento è entrato effettivamente a regime. L'obiettivo, più volte ricordato, è quello di promuovere i pagamenti *cashless* (ossia senza contante), al fine di introdurre l'abitudine all'utilizzo delle carte di credito ed evitare quindi fenomeni di evasione fiscale con i cosiddetti pagamenti in nero. Italia Viva ritiene che la digitalizzazione dei pagamenti sia un importante strumento di lotta all'evasione fiscale e in questo senso ci siamo mossi in precedenza con l'introduzione della fatturazione elettronica. È però indispensabile che si accerti che il *cashback* abbia effetti significativi sul gettito, perché la relazione tra l'uso del contante e l'evasione fiscale è piuttosto debole, così come al momento risulta incerta la direzione del nesso causale tra i due fenomeni. si tratta oggettivamente di un sistema che dovrebbe consentire di arrivare ai risultati di cui parlavo. Al contempo, non sfugge neanche la necessità di operare un bilanciamento tra interessi tutti meritevoli di tutela di tutela e che riguardi direttamente i costi e i benefici per una misura che comporta uno stanziamento cospicuo di risorse, eventualmente valutando anche strumenti che siano più utili e meno onerosi per favorire l'utilizzo della moneta elettronica (ciò, ovviamente, a fianco di questa iniziativa). Dai primi mesi di utilizzo di questo strumento si è dimostrato che l'operazione presenta però alcune criticità. Da taluni l'operazione è stata ritenuta eccessivamente onerosa ritenuta eccessivamente onerosa e ulteriori criticità sono emerse grazie alla segnalazione dei gestori delle stazioni di servizio e dei distributori, che hanno riferito dei cosiddetti furbetti di cui ha parlato il collega che mi ha preceduto in discussione generale. soggetti che, sfruttando alcune falle di questa misura, riescono a ottenere un maggiore rimborso, che permette loro di scalare rapidamente la classifica del superbonus *cashback*, aumentando le *chance* di raggiungere il premio di 3.000 euro l'anno. Il metodo più adoperato da tali soggetti è quello delle microtransazioni. Questo *modus operandi* consiste nel frazionare un unico acquisto in più transazioni. Sono operazioni assolutamente legali, ma che al contempo possono rappresentare costi eccessivi in termini di commissione per gli esercenti, i quali ovviamente sono obbligati, per ogni transazione, a pagare una commissione. Ovviamente, questo è un problema che andrà affrontato perché, per quanto minimo, comunque costituisce degli oneri a carico degli esercenti, come detto, e in qualche maniera bisognerà fare dei migliori controlli e trovare un sistema che

che si è registrato qualche giorno fa, nella Provincia di Siena, l'episodio in cui un soggetto, per pagare un rifornimento di carburante di 50 euro, ha fatto un numero incredibile di microtransazioni e l'operazione, per 50 euro di carburante, è durata 37 minuti. È evidente che il gestore del rifornitore avrà dovuto pagare per ogni minitransazione di uno o due euro la commissione e questo ovviamente incide molto carico, come dicevo, dei gestori e degli esercenti. Anche a fronte di tali criticità, quindi, si è manifestata più volte la volontà di utilizzare le risorse dello strumento anche per sostenere ristori e sostegni in questo delicato momento storico. Le ipotesi prospettate fino ad ora sono due: lo *stop* anticipato a tutto il programma *cashback* e cioè chiusura a luglio, così da salvare gli utenti che si sono registrati nel primo semestre e recuperare quindi tre miliardi, oppure la chiusura solo del super *cashback* (ogni sei mesi i primi 100.000 cittadini che fanno più transazioni ottengono 1.500 euro). Con il super *cashback*, quindi, è possibile guadagnare fino a 3.000 euro l'anno. In questo quadro, è più che mai necessario che le risorse messe a disposizione, che sono tutt'altro che illimitate, vengano utilizzate in canali che effettivamente possono far ripartire il Paese e che possono dunque agevolare le categorie più duramente colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica. Italia Viva - Partito Socialista Italiano ritiene invece che sia necessario procedere a una verifica approfondita sull'utilità di questo strumento e sulle sue criticità, così da poter apporre eventualmente i rimedi che sono necessari.

devono avere una messa a punto cammin facendo, per evitare quelle criticità di cui ho parlato in precedenza. È per questo motivo che Italia Viva - Partito Socialista Italiano voterà a favore dell'ordine del giorno per valutare i costi e i benefici concreti di questo strumento, in un quadro di intervento e di riforma, di modernizzazione e digitalizzazione dei pagamenti che sia il più ampio possibile, così da ottenere quei risultati che anche il *cashback* si proponeva di ottenere.

la mozione sul *cashback* che il Gruppo Fratelli d'Italia aveva presentato addirittura il 26 gennaio, per chiedere che i 5 miliardi buttati nell'inutile iniziativa del *cashback* e della lotteria degli scontrini fossero invece destinati a cose ben più utili, ad esempio a salvare imprese e posti di lavoro. L'avevamo presentata il 26 gennaio come Fratelli d'Italia, siamo stati molto felici quando le forze di centrodestra hanno chiesto di presentarla congiuntamente, cosicché la mozione che oggi discutiamo porta le firme non solo dei senatori di Fratelli d'Italia, ma anche quelle dei senatori della Lega e di Forza Italia. Grazie a questo la mozione presentata ha più di un quinto dei senatori come firmatari, quindi ha il privilegio di avvalersi della procedura abbreviata prevista dall'articolo 157 del Regolamento del Senato, che leggo testualmente perché, non essendo io il presidente Calderoli, non lo conosco a memoria: «Qualora una mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno della presentazione». Pertanto il Regolamento del Senato prevede

un Palazzo che se ne frega della legge per questioni ben più gravi come il Copasir e la tutela democratica delle istituzioni, figuriamoci quanto se ne può fregare dei Regolamenti del Senato. Tanto i vertici delle istituzioni, così come i grandi *media,* tacciono e la Corea del Nord è più vicina Giorgia Meloni, *leader* dell'opposizione democratica a questo Governo, ha scritto personalmente al *premier* Mario Draghi, per sottoporgli la questione del *cashback,* sapendo che lui almeno dedica maggiore attenzione a numeri e cifre. Ce lo immaginiamo, mani nei capelli, davanti a un faldone di numeri e calcolatrice alla mano. *Cashback*: 1.750 milioni di euro nel 2021, 3.000 milioni di euro nel 2022. Lotteria degli scontrini: 135 milioni di euro. Somma totale: 4.885 milioni di euro per *cashback* e lotteria degli scontrini, sottratti anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ve lo immaginate Draghi che deve giustificare questi importi in Europa? Non è facile, perché davanti a questa follia del *cashback* perfino

avere maggiore dignità. È possibile che nessuno Stato al mondo aveva avuto questa idea geniale della lotteria degli scontrini? Siamo andati a verificare e non è vero. L'Italia non è la prima; prima di noi lo Zimbabwe nel 2000 ha deciso, tramite la sua banca centrale, di introdurre una lotteria per cercare di favorire i consumi. La lotteria alla fine l'ha vinta il presidente Mugabe (quando si dice la fortuna),

la Banca centrale europea (BCE) nella lettera del 14 dicembre indirizzata all'allora ministro Gualtieri, ribadendo due concetti ricordati più volte. In primo luogo è non c'è un collegamento diretto tra uso del contante e lotta all'evasione. Lo afferma la BCE, ma lo ha anche detto, qualche tempo fa, l'allora ministro Padoan che, con tutto il rispetto per i colleghi del MoVimento 5 Stelle e per il collega che ha parlato prima di me, a occhio ne sa un po' più di loro di economia. Non c'è quindi collegamento tra lotta al contante e lotta all'evasione. Dove sta l'evasione? Nelle grandi multinazionali, nelle banche, nei negozi «apri e chiudi», cari ai cinesi, nelle cooperative fasulle, care alla sinistra, nei *money transfer* che il Governo ha detassato. Ecco, se volete fare la guerra all'evasione, secondo concetto, che la BCE ribadisce: il denaro contante, cioè la banconota di euro, è l'unica moneta a corso legale nell'eurozona. La moneta scritturale non è moneta a corso legale, è moneta privata in mano a istituti privati,

cara Corea del Nord non sarà attuato in Italia, non è nella facoltà dello Stato imporre a un privato la cifra cui deve vendere il suo prodotto. Le banche vendono quindi la loro moneta scritturale al prezzo che reputano più vantaggioso.

era questo il Governo più europeista della storia italica, da Enea in poi? E allora cercate, almeno su questo, di dare retta alla BCE. Pensate che noi di Fratelli d'Italia siamo talmente europeisti che chiediamo chiediamo che l'Italia abbia lo stesso limite al contante che ha l'economia che traina l'eurozona e cioè la Germania. Quest'ultima non ha limite al contante? Vorrà dire che non avremo limite al contante finché la Germania non ne porrà uno. A cosa serve incentivare la moneta elettronica? Semplicemente a favorire le banche e al Grande fratello

chi spende, per cosa. Noi pensiamo invece che un cittadino abbia la libertà di spendere il proprio denaro come meglio crede, senza doverlo spiegare a Governo e istituzioni. alla fine viene il sospetto che volete eliminare il denaro contante in modo da togliere le monete da 50 centesimi agli italiani per evitare che ve le tirino dietro quando uscite dal Palazzo.

gli aiuti dello Stato sono 11,3 a fondo perduto e 29 miliardi complessivi. A questo si aggiunge il cosiddetto decreto sostegni che mette in campo solamente 11 miliardi a fondo perduto. Questo vuol dire che le perdite complessive

un milione di posti di lavoro in meno; Confcommercio dice che 300.000 imprese sono a rischio e con loro due milioni di posti di lavoro. Davanti a tutto questo non c'è nessuno di buon senso che crede veramente che abbia una logica tenere 5 miliardi nel *cashback* e nella lotteria degli scontrini. A parole lo hanno già dichiarato tutti.

Fratelli d'Italia ha l'abitudine di far seguire i fatti alle parole che dice; ci auguriamo che le altre forze politiche abbiano la stessa decenza. Signor Presidente, l'Italia è in evidente e netto ritardo nella diffusione e nell'utilizzo della moneta elettronica: tutte le comparazioni internazionali. La media, in Italia, è di 61 transazioni con moneta elettronica per abitante, contro un dato europeo di 168 transazioni, per non parlare del Paese in in cui è più diffusa la moneta elettronica, la Danimarca, che è a quota 386, contro - lo ripeto - le 61 transazioni di un Paese come l'Italia, che invece è ai primi posti delle classifiche internazionali per diffusione della moneta contante, in rapporto al prodotto interno lordo, ovvero al volume dell'economia. Questo ritardo genera una serie di criticità, quali è il legame, dimostrato da numerosi studi, tra lo scarso utilizzo della moneta elettronica e l'ampiezza dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale, che è un problema strutturale del nostro Paese, quantificato in oltre 100 miliardi di euro dai rapporti che ogni anno vengono pubblicati in occasione della redazione della Nota di aggiornamento al DEF. C'è un secondo elemento di criticità, meno conosciuto, ma molto significativo, e sono i costi di gestione di questa enorme massa di contante presente nell'economia italiana, che la Banca d'Italia stima in miliardi di euro - credo si tratti di 8 miliardi di euro che ogni anno vengono bruciati per gestire i pagamenti in contanti, che invece potrebbero essere effettuati con strumenti più moderni, più sicuri ed enormemente meno costosi della gestione delle banconote e delle monete. Il precedente Governo Conte 2, ha varato un ambizioso piano di modernizzazione del nostro sistema di pagamento, il Piano Italia *cashless*. Il programma *cashback*, oggetto della mozione e dell'ordine del giorno

al 2022, ma è solo un pezzo, perché quel programma ha previsto anche l'abbassamento progressivo del limite di utilizzo della moneta contante, da 3.000 euro fino a 1.000 euro, il credito d'imposta a favore dei commercianti per i costi di gestione della moneta elettronica, la detraibilità di una serie di spese, solo se esse vengono effettuate con moneta elettronica, l'introduzione con un ammontare maggiorato del buono pasto elettronico, che passa da 7 a 8 euro, e la lotteria degli scontrini, che è diventata da poco operativa. Si tratta del programma più articolato tra quelli presenti a livello europeo. Il *cashback*, che è indubbiamente il cuore di questo programma, ha riscosso senza dubbio un notevole successo e di questo dobbiamo tenere conto, nel momento in cui ne andiamo a valutare i pro e i contro. Hanno attivato e si sono iscritti al programma oltre 8 milioni di cittadini, con 14.600.000 carte di pagamento e 355 milioni di transazioni registrate nel portale, che permette di accedere al programma. Una recente indagine, pubblicata dallo studio Ambrosetti, ci dice che quasi due terzi degli italiani giudicano favorevolmente questo programma di modernizzazione dei pagamenti, in particolare il programma *cashback*, e la stima dello studio Ambrosetti è di un potenziale di recupero del gettito fiscale fino a 4,2 miliardi di euro, a regime, per effetto dell'emersione

di questa ambizione ha bisogno di un sistematico monitoraggio, le cose da correggere sono via via emerse e sono state oggetto di un dibattito, che si è aperto nei mezzi d'informazione e a cui, nel mio piccolo, ho preso parte. La mia personale opinione che vadano introdotti elementi correttivi, una maggiore focalizzazione su alcuni elementi di questo programma, evitando che diventi regressivo, cioè che sia troppo generoso con persone ad alto reddito e non aiuti a evolvere verso la moneta elettronica - come è invece necessario - le fasce più deboli della popolazione. Credo che vada rafforzata la parte di aiuto e di sostegno nei confronti degli esercenti commerciali, che devono sostenere una serie di costi per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, come credo sia necessaria una riflessione costi-benefici sullo stanziamento di risorse per il programma *cashback*, perché 4,75 miliardi sono un ammontare molto consistente e lo sono ancora di più in una fase molto difficile dal punto di vista economico e sociale come quella che stiamo vivendo. Da questo punto di vista, credo che i contenuti che sono stati condivisi dalle forze di maggioranza vadano nella giusta direzione. Non è giusto, come è scritto nella mozione a firma Ciriani ed altri, sospendere il programma prima di aver fatto una valutazione rigorosa, numeri alla mano. Chiediamo questo al Governo: di fare una valutazione e mettere a conoscenza il Parlamento dell'andamento del programma e di intervenire con misure migliorative su un programma che sta dando un contributo, come ci dicono i primi dati

aiuterebbero il programma *cashback* a funzionare meglio, a fare fino in fondo il suo dovere di supporto alla modernizzazione del sistema dei pagamenti e ci permetterebbe cosa non disprezzabile - di risparmiare risorse significative rispetto allo stanziamento iniziale che potremmo destinare all'emergenza economica e sociale in una fase difficile per il Paese. Ritengo sia una posizione ragionevole: valutare e conoscere per poi deliberare, ed è per questo motivo che voteremo contro la mozione a firma Ciriani ed altri e sosterremo, invece, una diversa linea che ho cercato di esporre.

e purtroppo anche costantemente, molto preoccupanti. Cosa ci dicono? Ci parlano di una sottrazione di risorse importantissima, enorme per il Paese. Pensate voi cosa ciò significhi in questa pandemia,

e un costo economico, da ogni punto di vista. Capite soprattutto quali riflessi abbia l'utilizzo ampio del contante

sono molto chiari da questo punto di vista. Vi è stata un'adesione molto forte, ha ricevuto un forte gradimento da parte dei cittadini e ovviamente ha fatto sì che ci fosse finalmente un aumento enorme (da 9,6 milioni di

Come si fa davvero a non comprendere che è stato ed è uno strumento che ci ha fatto fare un grande passo in avanti nell'utilizzo dei pagamenti elettronici? Bisogna fare anche un altro lavoro, certo. Se infatti in Italia abbiamo un forte ritardo

Ma non credo assolutamente che dobbiamo criminalizzare o abbandonare questo strumento; dobbiamo invece monitorare e verificare se devono essere apportate delle modifiche per migliorarlo. Il *cashback* è uno strumento che si è dimostrato efficace e importante, e

all'ordine del giorno e il voto contrario alla mozione presentata da Fratelli d'Italia. signori del Governo, colleghe e colleghi, noi di Forza Italia non siamo mai stati innamorati della *bonus* *economy*, perché la riteniamo una politica economica che non premia veramente chi vale. Riconosciamo, come è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, che un certo beneficio c'è stato, ma attenzione: se abbiamo letto attentamente lo studio Ambrosetti, citato da qualche collega notiamo che questo sistema ha creato un ulteriore divario all'interno del Paese. È duplice, se volete: c'è un divario molto forte tra il Nord sviluppato, dove l'utilizzo del pagamento elettronico è più accentuato, ed altre parti del Paese che non lo hanno utilizzato; e, all'interno di questo, si è creata un'ulteriore distinzione: abbiamo visto che l'utilizzo del pagamento elettronico è favorito e utilizzato di più dalle persone che stanno meglio. Ecco, a noi una società che premia solo chi sta bene e non favorisce chi sta male non piace. Dobbiamo quindi favorire una crescita verso l'alto di tutti. ho sentito in discussione generale, tutti conosciamo la situazione attuale: oggi oltre ai *gap* infrastrutturali che hanno tanti nostri cittadini, per l'età e per la situazione economica, si è aggiunta anche la crisi da pandemia. Oggi, secondo me, questo strumento andrebbe attualizzato e verificato, perché riteniamo che siano cambiate un po' le cose da quando è stato concepito e messo in atto. Per avere una *community cashless society* servono dei pilastri e il *cashback* è uno di questi; non ha senso pensare di poter recuperare quel *gap* che è stato richiamato fermandoci solo al *cashback*. Serve una visione strategica, ambiziosa e sistemica per la *cashless society* in Italia, ma non l'abbiamo; ci siamo fermati solo alla prima fase. È vero che in valore assoluto le percentuali sono state minime, ma nell'opinione pubblica hanno dato molto fastidio i furbetti che andavano a fare 10 centesimi di benzina per poter entrare nella lotteria. Una società che punta sulla lotteria a noi non piace; ci piace di più una società più concreta. *(Applausi)*. Vogliamo anche ricordare che nel nostro ordine del giorno è scritto dobbiamo tarare e aggiornare la situazione, creare un tavolo di concertazione e di verifica puntuale, per vedere se gli strumenti messi in campo siano stati realizzati e rispondano in pieno alla visione che avevamo prima.

Non dobbiamo farne una battaglia ideologica, ma dobbiamo concentrarci sulle cose che effettivamente e realmente servono. È chiaro che c'è tutto un mondo che sta nascendo e che ruota attorno alla *cashless society*, attenzione perché i *gap* che dobbiamo recuperare nel nostro Paese sono molteplici e andare avanti solo sul *cashback* vuol dire fare solo una piccola parte di *step* successivi che al momento non siamo in grado di fare. Le condizioni sono cambiate; il concerto macroeconomico è cambiato; la pandemia ha avuto delle varianti inattese che stanno aggravando ancor più la nostra economia. Abbiamo visto cosa

dalla ragione al torto se trasformiamo atti di legittima e democratica protesta in atti di violenza. Esprimiamo, pertanto, solidarietà alla Polizia e alle Forze dell'ordine che preservano l'ordine democratico nel nostro Paese.

dall'Osservatorio sulla spesa pubblica, che dava dei numeri diversi. Prendo atto di quanto che lei ha detto e andrò a verificare. È evidente che, essendo *bonus*,

reale. Io direi di no alla fine oggi. Tariamoci; verifichiamo il punto esatto della situazione e, una volta condivisa - spero - dalla maggioranza più ampia possibile all'interno del Parlamento, possiamo ripartire.

particolarmente ben fatta. A me non piace essere ipocrita e, quindi, partiamo da questo presupposto. Giustamente la senatrice De Petris è intervenuta dicendo che è giusto monitorarlo, così si va avanti in quella direzione, ma io posso dire che dal punto di vista della Lega, in realtà, il monitoraggio deve servire per far sì che la manovra venga corretta e che il *cashback* possa essere anche evidentemente eliminato, se proprio non funziona bene.

presentata da Fratelli d'Italia sull'abolizione del *cashback*. Qualcuno potrebbe allora chiedere: perché voi della Lega, ma anche i colleghi di Forza Italia, avete sottoscritto questo ordine del giorno, che dice tutto e il contrario di tutto?

lavora in una cornice europeista. Così ci è stato detto, visto che qualcuno addirittura ci ha fatto notare che ci siamo convertiti all'europeismo. Bene, se lavoriamo nella cornice europeista, dobbiamo fare quello che l'Europa ci dice di fare su questo tema. Giusto? Allora, io sono certo che il presidente Draghi non potrà non tener conto delle osservazioni che la Banca centrale europea ha fatto al Governo italiano, scrivendo una letterina indirizzata al gentile Ministro. È una letterina che dice che dovrebbe sussistere una chiara prova che il meccanismo di *cashback* consente di conseguire la finalità pubblica nella lotta all'evasione fiscale. La letterina dice che il rimborso speciale di 1.500 euro sembra essere progettato per incentivare l'uso di pagamenti elettronici per importi limitati, che potrebbero essere, invece, pagati in moneta. Dovrebbe, inoltre, tenersi presente che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, per varie e legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante, altresì generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, è rapido ed agevola il controllo sulla spesa di chi paga. In aggiunta, i pagamenti in contanti non richiedono una infrastruttura tecnica funzionale e relativi investimenti e sono sempre disponibili. Ciò riveste particolare importanza in caso di un'interruzione della corrente elettrica, che rende i pagamenti elettronici indisponibili. infine, i pagamenti in contanti agevolano l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia, consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria. In questo contesto, la BCE ritiene che l'introduzione di un programma *cashback* per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata, alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti, in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili. La BCE apprezzerebbe, La BCE apprezzerebbe, ovviamente nei confronti di un Governo super europeista, che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono, adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la Banca centrale europea, se del caso. Quindi, ce lo chiede l'Europa e siamo certi che il presidente Draghi, dopo un bel monitoraggio, capirà che questa norma non funziona e non va bene. Non perché siamo degli ipocriti, ma perché sappiamo bene come vanno le cose. Di conseguenza, perché non dovremmo fidarci del presidente Draghi? Questa è la nostra scelta. Così almeno l'avete capito anche voi: ne sono contento e mi fa piacere. Inoltre, sono stati spesi 4,75 dei 10 miliardi destinati alla digitalizzazione, quel programma previsto nel Piano di resistenza e resilienza,

che, a detta di tutti, deve essere l'elemento portante per la rinascita del nostro Paese, favorendo l'economia, le aziende e il rapporto con i cittadini. Se si una cifra così cospicua da quella linea di intervento, non penso che l'Europa sia molto contenta e molto soddisfatta di questo. C'è da dire che, in certi casi, non solo siamo europeisti, ma ci mettiamo anche in stato di adorazione nei confronti di questo europeismo, che fa capire e comprendere bene che certe cose che facciamo non sono assolutamente buone e vanno assolutamente riviste. Concludo, sperando di non usare tutto

che si apprestano a seguire le indicazioni che diamo loro; ce l'ho con qualcun altro, se non fosse ancora chiaro. Guardiamo cosa succede in Finlandia, dove nel 2018 cento dei pagamenti totali è stato effettuato con le carte di credito o di debito o con le *app*, mentre l'uso del denaro contante si è ridotto al 19 per cento.

che è una cosa normale e di buon senso. Se pago in contanti, mi rendo conto di quello che sto pagando; con la carta di credito e con il bancomat, invece, non è che segno e ho tutto sotto controllo. È una cosa normale. Ma allora noi dobbiamo fare qualcosa

dotato di grande pragmatismo e di grande attenzione, saprà farsi valere su questo punto, rispettando le indicazioni dell'Europa, tutelando i cittadini da eventuali ulteriori debiti e, d'altra parte, proponendo misure di contrasto all'evasione fiscale più serie,

Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, oggi siamo qui a impegnare il nostro tempo per discutere di una mozione che dimostra la più totale miopia politica. Prima di spiegare perché il *cashback* è una misura fondamentale, vorrei attraversare alcuni punti della mozione, perché è quel documento che pone sotto accusa il *cashback*; quindi è opportuno analizzare quel che c'è scritto, prima di passare a spiegare perché invece è buona cosa continuare con la misura.

fin qui hanno detto una cosa giusta, perché il *cashback* serve per aumentare il tasso di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani ed è quello che sta riuscendo a fare.

mesi. La mozione prosegue dicendo che il *cashback* è la misura più nota del Piano Italia *cashless*. È vero, ma qui la vera notizia è che il *cashback* è parte di un piano ben più ampio, che è quello, appunto, di portare l'Italia verso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, in linea con gli altri Paesi, dove utilizzare la plastica - così si dice in gergo - è cosa normale anche per il pacco di caramelle e questo ormai da tempo immemorabile. Dobbiamo ricordare che l'Italia - qualcun altro l'ha già detto - è un'economia *cash-based* fra le trentacinque peggiori al mondo, secondo il *cash intensity index*, che è un indice che misura l'incidenza del contante sul PIL. Per quanto invece riguarda il *cashless society index* è al ventitreesimo posto nell'Unione europea. La mozione prosegue attingendo a piene mani dalla lettera inviata all'allora ministro Gualtieri da parte di Yves Mersch,

Ora, non so quante delle persone qui presenti e quanti degli 82 firmatari della mozione abbiano letto integralmente quella lettera e non solo le parti riportate dai giornali, ma questa lettera è un coacervo di indicazioni, spesso arzigogolate, che concludono con un semplice rilievo all'Italia per non aver avvisato la BCE prima di porre in essere l'iniziativa del *cashback*. qualcosa che però mai mi sarei aspettato venisse eccepito da Gruppi politici cosiddetti sovranisti presenti in questo Senato, che oggi si definiscono europeisti, patriotticamente europei.

e ancora che l'Unione non affronta «esplicitamente la questione se, o in quale misura, sia consentito introdurre una restrizione di ordine più generale all'obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro». Ma dove mai è inserita nel *cashback* questa restrizione? Da nessuna parte. E poi si dice che qualunque limitazione o disincentivo diretto o indiretto ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro; ma qui non si parla di incentivo, si parla di disincentivo. E la cosa non è la stessa, perché a seconda di come viene riportata e utilizzata da stampa o Gruppi politici, assume caratteri diversi. Secondo Mersch non si può incentivare qualcuno a fare qualcosa per modificare i comportamenti e le politiche della Nazione. Allora, se questa è la logica, aboliamo direttamente tutti gli incentivi previsti per le imprese, perché così dovremmo fare secondo lui. Poi Mersch scrive ancora (ed è sempre una parte riportata nella mozione, come ha detto anche prima il senatore Romeo): «la BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l'evasione fiscale» - e qua ci ritorno «può, in linea generale, costituire un "interesse pubblico" che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell'uso dei pagamenti in contanti». In pratica, nella stessa lettera ritorna sui suoi passi, cioè dice che si potrebbe anche fare. Però qui c'è un appunto da fare a beneficio di chi ci segue, ma soprattutto di coloro i quali hanno scritto questa mozione, perché l'hanno costruita incentrandola sulla lotta all'evasione fiscale che per loro è il perno del *cashback*. Quando il MEF ha inviato ad ottobre 2020 il regolamento del testo in esame, oltre a tutte le varie indicazioni (relazione tecnica, analisi tecnico-normativa), ha inviato anche l'Analisi dell'impatto della regolarizzazione, la cosiddetta AIR, che dice che, in linea di principio, la nuova disciplina avrà un impatto sistemico importante in termini di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici da un lato, di trasparenza e tracciabilità delle transazioni in denaro dall'altro. Si prevedono effetti diretti positivi sulla finanza pubblica in termini di diminuzione del costo del denaro contante e - attenzione potenzialmente di riduzione e contrasto all'economia sommersa. Su quattro parametri, il quarto è quello della riduzione dell'economia sommersa e si dice anche «potenzialmente»: quindi è qualcosa di non ricercato, né quantificato. Quindi, ridurre il *cashback* a una misura per la lotta all'evasione fiscale significa non aver compreso la misura stessa. Ma siamo qui per spiegare e far capire se il *cashback* ha raggiunto gli altri obiettivi, ossia i primi tre. Di certo gli operatori bancari ultimamente hanno rilasciato un po' di indicazioni. Chi utilizza la carta di credito e aderisce al *cashback* la usa il 22 per cento in più di chi ha la carta di credito in tasca ma non aderisce

Ciò significa che sono aumentate le transazioni e, quindi, la spesa verso i piccoli commercianti, che sono proprio coloro che dobbiamo cercare di supportare con un rilancio dell'economia e non solo con il ristoro di quanto perso.

affermando che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni (non dice quali e sorvoliamo sul perché),

probabilmente letto bene il documento perché si è incentrata solo sull'aspetto fiscale, che - ripeto - è al quarto punto. Quindi è favoloso il commissario Mersch che alla fine fine ci dice qual è il punto di passaggio dalla convenienza nell'utilizzo del contante alla plastica. Lo dice lui e senza neanche aver verificato le motivazioni.

tutte quelle attività costrette alle chiusure, in quanto tutelare il lavoro è un dovere dello Stato, così come lavorare è un diritto del cittadino. In realtà, non avete fatto altro che confermare che il *cashback* è un'ottima misura, in quanto supporta proprio il rilancio di tutti quegli operatori che oggi, con il solo ristoro, non farebbero altro che coprire parte dei costi sostenuti, mentre con anche il *cashback* si genera una spesa aggiuntiva che li aiuterà a ritornare a una vita normale. *(Applausi)*. E sappiamo benissimo che, in questo periodo, il risparmio in Italia è cresciuto proprio perché non si spendeva. L'applicazione IO, su cui si basa il sistema gestito da PagoPA, è una soluzione innovativa che amplia le possibilità per i cittadini, le imprese e gli enti locali. Più i cittadini saranno presenti su quest'applicazione, più i Comuni potranno fornire servizi in modalità totalmente nuova, a vantaggio delle necessità del Comune stesso e dei cittadini. Tra l'altro - lo ricordo un po' per tutti - nel PNRR abbiamo inserito anche il concetto di fisco in un'*app* proprio per migliorare il rapporto fra Agenzia delle entrate e cittadini, semplificando l'accesso al fisco

Certo, come per ogni misura, dopo un periodo di applicazione, è sicuramente corretto verificare i parametri e i risultati e capire se è necessario orientare meglio gli sforzi in una direzione o in un'altra al fine di massimizzare i risultati. E sebbene abbia senso pensare di farlo

la mozione che abbiamo presentato come Gruppo Lega parte dal presupposto, trattandosi di un argomento di grande attualità,

C'è un dibattito aperto sul tema da diverse settimane. Sono diversi i medici che

che - è stato verificato - sono riusciti a evitare l'ospedalizzazione dei pazienti curandoli direttamente a domicilio.

che si tratta di Covid, magari ancora prima del risultato del tampone e, quindi, prescrivono subito degli antinfiammatori. E questo sistema di utilizzo rapido curare subito il paziente riesce a fermare la malattia e a evitare che possa degenerare in un qualcosa di molto grave che costringe ad andare in ospedale. Abbiamo illustri persone che hanno rilasciato diverse interviste sui giornali, dal professore Remuzzi, al dottor Mangiagalli, al dottor Cavanna. Ci sono esperienze dirette di questi medici a tal proposito desidero ringraziare il sottosegretario Sileri perché ha ricevuto questi medici che si sono riuniti e hanno organizzato anche dei comitati.

e ascoltato le loro richieste e oggi siamo qui a cercare di prendere tutti insieme un impegno politico affinché il Ministero della salute

sul protocollo, in modo tale che si possa poi agire in maniera più decisa e, quindi, prendiamo esempio da tutte le esperienze. Io penso che questo sia il metodo migliore. Il Sottosegretario ha già dato disponibilità, ma, giustamente, diamo anche un segnale politico forte, a tutta la comunità nazionale, che ci stiamo occupando del tema. E, sono convinto che il lavoro proseguirà in questa direzione. Visto, poi, che si è anche trovato un ordine del giorno comune, annuncio già

colleghe e colleghi, l'ultimo anno ha cambiato le nostre vite per sempre e ha cambiato il nostro modo di guardare al Sistema sanitario nazionale. Sono entrati in uso comune termini che mai avremmo immaginato di conoscere. Sappiamo tutto - per esempio di test antigenici, molecolari, indici di contagio Rt. Il SARS-Cov-2 è entrato nelle nostre vite stressando la capacità di risposta delle strutture sanitarie e ci ha fatto capire che la precoce individuazione dei casi, la rapidità dei test diagnostici, la permanenza a domicilio per quarantena o isolamento dipendono fortemente dall'organizzazione territoriale presente nei diversi contesti regionali. E qui ci sarebbe molto da dire. dire. Pertanto, è necessario rafforzare la rete dei servizi territoriali per ridurre la necessità di ricovero ospedaliero e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari ospedalieri. Ancora oggi sentiamo di situazioni di difficoltà nel garantire l'assistenza territoriale a tutte le persone che necessitano di percorsi diagnostici e terapeutici connesse all'emergenza Covid-19; nel fornire indicazioni operative volte ad identificare e prendere in carico precocemente i pazienti con sospetto Covid-19; nel garantire la sorveglianza sanitaria e assistenza alle persone fragili, in quanto più esposte a rischio e alla necessità, anzi, di un implementata presa in carico Stiamo procedendo sempre più speditamente con la campagna vaccinale, ma non dobbiamo trascurare i tanti che ancora oggi contraggono il virus. Il trattamento precoce delle infezioni ha valenza preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e sub-intensiva. Quindi, bisogna favorire le terapie domiciliari precoci e l'utilizzo di anticorpi monoclonali, che finalmente sono disponibili nel nostro Paese anche grazie all'impegno della mia collega Castellone e del sottosegretario Sileri. Inoltre, bisogna garantire la presa in carico territoriale delle persone dimesse da ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l'obiettivo di migliorarne l'appropriatezza, offrendo assistenza alle persone ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio; un percorso che poi deve diventare e restare uno dei pilastri di un rinnovato sistema sanitario, come diciamo da tempo. Purtroppo, affrontare la pandemia ha comportato anche la riduzione delle attività ordinarie e una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto di quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica che assume particolare rilevanza nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Per queste ragioni, con la nostra mozione chiediamo che siano aggiornati protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici del territorio dei pazienti Covid-19; che sia istituito un tavolo di monitoraggio ministeriale in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale. Insomma, come diciamo da sempre, l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale, la telemedicina sono punti fondamentali per migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza lo abbiamo evidenziato e abbiamo chiesto che si punti davvero su una medicina incentrata sul paziente e i suoi bisogni, sulla persona e non sulla malattia. Oggi chiediamo la stessa cosa. I malati Covid-19 devono essere assistiti nel migliore dei modi già nelle loro case, perché solo intervenendo in tempo e nel modo più giusto riusciremo a diminuire e scongiurare il peggioramento della malattia, con il successivo e drammatico ingresso in terapia intensiva. *(Applausi)*. Solo così riusciremo ad alleggerire i nostri ospedali e pian piano, complici i vaccini, a tornare gradualmente alla socialità, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista sanitario, economico e anche umano. Inoltre, come ha annunciato precedentemente il senatore Romeo, anche noi procederemo a ritirare la nostra mozione per convergere sull'ordine del giorno che abbiamo tutti firmato. Dichiaro aperta la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà. Signor Sottosegretario, la ringrazio dell'attenzione e ringrazio anche ai colleghi che hanno presentato le mozioni in esame e hanno permesso di fare un lavoro comune, insieme, per arrivare a una soluzione condivisa su un tema che nell'ultimo anno abbiamo affrontato già più e più volte e che ci ha visto interrogarci sul nostro Sistema sanitario nazionale, soprattutto per quanto

- è stato ben sottolineato che nell'ultimo anno ci siamo trovati davanti a una malattia sconosciuta. La medicina non è una scienza esatta,

Questo ha fatto sì - lo sappiamo tutti, ma la memoria è importante - che gli ospedali si siano trovati sovraccarichi. E purtroppo questo è un fatto che verifichiamo anche in questi giorni - ahinoi - perché la situazione non è cambiata molto.

curare le persone e non intasare gli ospedali. È fondamentale, come chiede la mozione, un aggiornamento costante e continuo delle linee guida, in modo che la somministrazione dei farmaci più efficaci e la presa in carico del paziente possano avvenire nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. In questo è essenziale la figura del medico di medicina generale, dei pediatri e di tutti gli specialisti che a livello territoriale hanno a che fare con le persone. Guardate, colleghi, questo è fondamentale per due motivi: non soltanto per dare una cura pronta a chi si ammala, ma anche per sostenerlo, perché i medici di medicina generale il più delle volte conoscono la situazione, anche familiare e sociale, in cui il malato vive. Sappiamo ormai essere molto importante e

che fossero efficaci ed efficienti. La sorveglianza sanitaria è fondamentale nel nostro sistema per garantire la salute nel miglior modo possibile e anche un'assistenza - come diceva la collega prima di me

abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno e crediamo davvero che i territori che meglio hanno affrontato la situazione possano essere di esempio per altri territori che ancora lottano con criticità davvero notevoli. Speriamo che da qui in avanti il nostro sistema sanitario a livello territoriale possa migliorare, non soltanto per questa emergenza, ma anche per tutte le altre situazioni giornaliere che si troveranno ad affrontare. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Sottosegretario, sono gravi le ripercussioni che la pandemia ha avuto sul servizio sanitario in poco più di un anno: si sono registrati oltre 3 milioni e mezzo di casi, con oltre 111.000 morti. Ancora oggi risultano ricoverati circa 30.000 pazienti Covid e le terapie intensive in molte Regioni sono sopra la soglia di sicurezza. In Italia, stando ai più recenti studi, è aumentata del 40 per cento la rinuncia alle cure dei pazienti non Covid, con oltre due milioni di *screening* oncologici in meno e 13.000 diagnosi diagnosi di malattie mancate. Questo comporta non soltanto un danno diretto a chi non ha potuto curarsi al momento giusto in maniera adeguata, ma anche un danno indiretto al Servizio sanitario nazionale in termini di costi e gestione. In effetti, il nostro Servizio sanitario nazionale dovrà assistere

oltre che creare più sofferenza al malato, comporta l'utilizzo di terapie più complesse e spesso invasive. Gli ospedali sono stati sovraccaricati di lavoro per il Covid-19 e hanno dovuto limitare di molto l'accesso alle cure dei pazienti non Covid, che avevano bisogno di assistenza ospedaliera. In effetti, molti reparti sono stati chiusi per essere riconvertiti in reparti Covid e le terapie intensive, dal numero limitato, sono state utilizzate per i casi Covid più gravi, non permettendo l'utilizzo per il fabbisogno salute del Paese legato ad altre patologie non meno gravi. Le mozioni oggi in discussione perseguono il duplice meritorio obiettivo di fornire cure adeguate ai malati Covid, quando gli stessi si trovano presso la propria abitazione, ed evitare sia l'ospedalizzazione, sia i conseguenti problemi di sovraffollamento delle strutture sanitarie, che - come abbiamo anticipato - vanno in sofferenza quando il carico di malati si intensifica a causa dell'andamento della curva dei contagi. Il nostro Gruppo, Forza Italia, ha sempre sostenuto quanto previsto dalle mozioni in discussione oggi in Aula, ribadendo da sempre l'importanza del potenziamento della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con le eventuali unità di assistenza presenti sul territorio. Cogliamo anche questa occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari, tutti i medici e tutti coloro che ogni giorno prestano assistenza Ci sentiamo di condividere la necessità che la cosiddetta «vigile attesa», prevista nella circolare ministeriale e nelle raccomandazioni AIFA, che consiste di fatto in un'osservazione degli eventuali miglioramenti o peggioramenti di un malato Covid presso le rispettive abitazioni, sia rivisitata in un concetto più dinamico e non solo statico, come oggi è interpretata, così da consentire che, grazie al supporto medico, i casi con sintomatologia lieve restino tali e i casi che invece possono aggravarsi non si aggravino. Della mozione condividiamo anche la proposta di istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo. Condividiamo anche la necessità di definire, per il tramite di AIFA, protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid e l'opportunità di ricorrere alla somministrazione preventiva a pazienti paucisintomatici con tampone positivo delle terapie antivirali e di prevenzione delle complicanze polmonari in fase sperimentale e *off label* secondo protocolli già in uso, ovvero in esito alla rilevazione di evidenze di efficacia nazionale e internazionale nell'ambito del *trial* in essere. Abbiamo proposto l'obbligatorietà del vaccino per medici e operatori sanitari al fine di rendere più sicuri i luoghi dove si dà assistenza sanitaria ai malati. Abbiamo proposto lo scudo penale ai vaccinatori per incentivare il reclutamento di operatori che inoculano il vaccino. Abbiamo promosso la vaccinazione nelle farmacie per rendere più accessibile e capillare la vaccinazione. stato e sarà sempre quello di sostenere il Paese e supportare gli italiani tutti (dai più piccoli ai più grandi, da chi non lavora, alle imprese in crisi, da chi soffre il disagio sociale a chi è

di poter resistere in questo difficile momento che attraversa l'umanità, in attesa che arrivi la luce per tutti. Forza Italia c'è e sarà sempre a fianco degli italiani. Signor Presidente, ogniqualvolta me ne viene data occasione ripeto che sono molto importanti le risorse e adesso, con i fondi europei, (non solo a PNRR), le risorse ci sono anche per innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto al Covid, partendo dall'analisi del rischio genetico e la relativa risposta individuale al virus, tra l'altro oggetto di un vasto studio della comunità scientifica internazionale di cui fanno parte anche numerosi scienziati italiani,

La presa in carico appropriata e tempestiva del paziente a domicilio, quanto mai necessaria in emergenza Covid, è il terreno in cui oggi ci troviamo a misurarci. Bisogna essere sufficientemente flessibili per cogliere tutte le innovazioni che hanno un supporto scientifico

validati tali da essere giustificabili come risposte solide e rigorose alla malattia, senza rischi di dare tossicità ai pazienti e la finalità ultima della nostra mozione, coerentemente a quanto è stato poi dedotto nell'ordine del giorno, è quella di impegnare il Governo a una sensibilizzazione che ne tenga debito conto, facendo valore aggiunto delle migliori esperienze cliniche conoscenze scientifiche, dando prova di efficienza e appropriatezza, investendo in prevenzione, medicina predittiva, personalizzazione delle cure, verifiche rigorose, sostanziali e mirate in aggiornamento e monitoraggio continuo. Noi siamo tra coloro che intendono ridisegnare l'Italia con una visione, la visione della sanità sostenibile del futuro, di tutela universalistica della persona e della famiglia, prima ancora o comunque al sorgere della malattia, consapevoli che le risorse del PNRR, in quanto *one shot* e quindi irripetibili, devono essere utilizzate solo per processi migliorativi che consentano da subito di dare di più costando di meno, implementando vera integrazione tra rete ospedaliera e territorio, con domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure da remoto, secondo protocolli nazionali definiti *in progress*,

Il governo della pandemia è prevenzione e cura precoce, limitando l'ospedalizzazione ai soli casi proattivamente eleggibili: l'azzeramento del sovraccarico evitabile di ospedali e terapie intensive con un'immunizzazione di massa delle categorie fragili è precondizione per il ritorno alla normalità, una sfida alla normalità, una sfida possibile a cui questa maggioranza può rispondere al servizio del Paese, agendo in potenziamento e capillarizzazione della sorveglianza attiva e genomica del virus e delle sue varianti, in profilassi vaccinale selettiva e cure domiciliari aggiornate tempestivamente ed evolutivamente in ragione delle

Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghe e colleghi, le mozioni in discussione oggi affrontano la fondamentale tematica delle cure domiciliari, nello specifico il loro necessario potenziamento in riferimento al trattamento sanitario dei pazienti affetti da Covid-19. Entrambe sono fortemente condivisibili, perché toccano una materia verso la quale questa legislatura è fortemente impegnata da anni e ancora prima del tragico avvento della pandemia da Covid-19. Covid-19. Le cure domiciliari, infatti, e più in generale il tema dell'assistenza territoriale sono gli aspetti che dimostravano e dimostrano tuttora le maggiori carenze in ambito sanitario del Servizio sanitario nazionale e la diretta conseguenza di queste carenze è storicamente rappresentata dall'intasamento dei nostri ospedali, con una intollerabile diminuzione riscontrata nella qualità del servizio offerto ai pazienti, specialmente quelli fragili e bisognosi di cure adeguate. Cito, a titolo esemplificativo, anche per mia diretta esperienza professionale, il sovraccarico dei pronto soccorso in tutta Italia: troppe volte, infatti, nella mia trentennale esperienza di medico di pronto soccorso, ho assistito all'arrivo di pazienti che non necessitavano del ricovero, ma che in mancanza proprio di un'adeguata assistenza territoriale domiciliare arrivavano in ospedale convinti che il ricovero potesse rappresentare la migliore soluzione per il loro stato di salute. Al contrario, l'intasamento degli ospedali ha purtroppo causato un effettivo rischio per il paziente, ovviamente a livello sanitario, anche per eventuali infezioni nosocomiali, ma anche a livello psicologico, perché un ricovero rappresenta un evidente stress con dirette conseguenze negative. Le cure domiciliari, invece, laddove valutate come opportune dal medico curante, insieme al fondamentale ausilio della telemedicina, possono sicuramente contribuire a un positivo decorso del paziente, eliminando peraltro il ricorso all'ospedalizzazione contribuendo al benessere complessivo della persona coinvolta e degli eventuali familiari. La sfida che abbiamo raccolto in questa legislatura è stata, quindi, di intervenire su questi mali ormai cronici del nostro Servizio sanitario nazionale, evidentemente frutto di una perversa logica centrata sulla inevitabile ospedalizzazione, anche quando la cartella clinica del paziente non motivava fino in fondo questa scelta, che dovrebbe altresì rappresentare l'ultima soluzione sanitaria. provvedimenti sono stati già adottati: penso, *in primis,* alla figura dell'infermiere di famiglia, con il cosiddetto decreto rilancio, vera svolta per la medicina territoriale, in una logica positiva di sinergia con tutti gli altri livelli di assistenza sanitaria. Con lo stesso provvedimento sono stati previsti importanti finanziamenti per l'assunzione di migliaia di infermieri; adesso tocca alle Regioni adottare velocemente ogni provvedimento utile

per l'instancabile impegno durante la pandemia - dovrà essere stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli infermieri del servizio di emergenza territoriale 118 saranno assunti mediante procedure concorsuali pubbliche e dovranno possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Per i mezzi mobili di soccorso del servizio di emergenza territoriale, il 118 si dovrà avvalere di personale adeguatamente formato con dei corsi teorico-pratici per le funzioni di autista e soccorritore, altra importantissima figura verso la quale evidenzio ancora una volta l'opportunità di arrivare finalmente a un doveroso riconoscimento giuridico. Da tutti questi elementi, che in questa sede brevemente ho sottolineato, risulta evidente il concreto lavoro istituzionale che si sta svolgendo in tema di assistenza territoriale e cure domiciliari. Le mozioni oggi in esame vanno pienamente in questa direzione. A loro va il mio convinto appoggio nell'ottica di un complessivo miglioramento del nostro Servizio sanitario nazionale, verso il quale continueremo a impegnarci con l'adozione di altri e fondamentali provvedimenti.

Avverto che le mozioni sono state ritirate e sono stati presentati l'ordine del giorno G1, a firma del senatore Ciampolillo, e l'ordine del giorno G2, a firma dei senatori Romeo, Castellone, Binetti, Errani, Boldrini, Zaffini, Parente e di altri

Senatore Ciampolillo, se permette al Sottosegretario di dare il parere sugli ordini del giorno, il suo intervento sarà anche più sostenuto dal parere del Sottosegretario.

di ribadire ciò che è stato fatto e ciò che deve essere fatto per le terapie domiciliari dei pazienti affetti da SARS-Cov-2. Cercherò di essere molto breve. L'infezione da SARS-Cov-2 è una condizione estremamente complessa. Abbiamo iniziato a conoscerla nel dicembre 2019 abbiamo imparato a conoscere meglio il virus durante la prima ondata, purtroppo durante la seconda e ora che stiamo vivendo la terza. Vi sono meccanismi fisiopatogenetici molto complessi, connessi per la molteplicità delle manifestazioni cliniche e per il ruolo rivestito dalla risposta immunitaria particolare dei singoli soggetti. Le terapie si sono evolute nel tempo e a tutt'oggi non sono completamente chiare. Vi sono moltissimi protocolli ancora in essere; non parlo solamente dell'Italia, ma del pianeta intero. Abbiamo accumulato informazioni relative alla patogenesi della condizione morbosa e ai sintomi presentati dai pazienti; abbiamo imparato, soprattutto nelle fasi iniziali, che vi erano sintomi inizialmente inizialmente sottovalutati e poi successivamente più noti. Successivamente si sono via via acquisite conoscenze nell'ambito dell'efficacia e della tossicità correlate alle differenti terapie adottate. In particolare, il trattamento terapeutico della patologia si è articolato su diversi approcci differenziati, che sono andati a coinvolgere *in primis* farmaci a potenziale attività antivirale contro il SARS-Cov-2, farmaci ad attività profilattica e terapeutica contro le manifestazioni trombotiche, farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria e infusioni di plasma mirate a un trasferimento di anticorpi neutralizzanti il legame tra il nuovo coronavirus e il suo recettore espresso dalle cellule umane. È opportuno sottolineare che ancora oggi esistono larghi margini di incertezza rispetto all'efficacia di alcuni degli approcci terapeutici appena menzionati e che l'uso delle differenti terapie piuttosto che l'assenza di impiego delle stesse dipendono dalla severità delle manifestazioni cliniche presentate dai malati. Proprio in considerazione dell'alto livello di incertezza con cui queste terapie sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza rispetto a una pandemia che in effetti stiamo imparando a conoscere - come ho detto prima - giorno per giorno, è importante aggiornare continuamente le informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza che si rendono progressivamente sempre più disponibili. A tale scopo, la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA ha predisposto una serie di schede che rendono espliciti gli indirizzi terapeutici entro cui è possibile prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci utilizzati nell'ambito di questa grave emergenza. Le schede riportano in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza ad oggi disponibili, nonché le interazioni e le modalità d'uso raccomandabili nei pazienti con Covid-19. Nello stesso formato vengono individuati i farmaci per cui è bene che l'utilizzo rimanga all'interno di sperimentazioni cliniche controllate. In data 30 novembre 2020 è stata adottata la circolare del Ministero della salute n. 24970 in merito alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da SARS-Cov-2, al fine di fornire adeguate indicazioni operative, tenuto conto dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale. In tale circolare viene segnalata la necessità di razionalizzare le risorse al fine di poter garantire la giusta assistenza a ogni singolo cittadino in maniera commisurata al grado e alla gravità del quadro clinico. La circolare riporta, tra l'altro, che i National Institutes of Health statunitensi hanno formulato una classificazione fondata anche sui criteri radiologici e con i limiti e le difficoltà legate alla realizzazione di questa indagine in una situazione pandemica in cui vengono individuati cinque stadi clinici della malattia. Nel paragrafo "Principi di gestione della terapia farmacologica" viene specificato che le indicazioni fornite si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di Covid-19. viene sottolineato che, onde evitare il rischio di ospedalizzazioni tardive, nel caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente durante la fase di monitoraggio domiciliare, andrà eseguita una rapida e puntuale rivalutazione generale per verificare la necessità di un'ospedalizzazione o di una valutazione specialistica del soggetto. Nella medesima circolare è stata altresì delineata una rappresentazione schematica del monitoraggio del soggetto infettato da SARS-Cov-2 e della dinamica possibilità di transizione da paziente a basso rischio a paziente con quadro in evoluzione peggiorativa, tale da richiedere o una modifica della terapia o un ricovero un ricovero ospedaliero. Le raccomandazioni fornite dalla circolare riflettono i dati della letteratura scientifica e tutte le informazioni attualmente esistenti. I trattamenti sintomatici, come il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista una chiara controindicazione all'uso. Altri farmaci sintomatici possono essere utilizzati in base al giudizio clinico. Non esistono infatti ad oggi evidenze solide e incontrovertibili, ovvero derivanti da studi clinici controllati, di efficacia e sicurezza per l'impiego di altre terapie nelle prime fasi della patologia in questione. Un esempio su tutti può essere l'indicazione a non utilizzare routinariamente i corticosteroidi. Tale raccomandazione si basa sul fatto che attualmente esistono evidenze di un beneficio clinico di tali farmaci solo in questo *setting* di pazienti/fase di malattia. È necessario ricordare che in molti soggetti con malattie croniche l'utilizzo del cortisone può determinare importanti eventi avversi che rischiano di complicare il decorso della malattia virale. Sono stati resi disponibili per le terapie anti Covid-19, con il decreto del Ministero della salute del 6 febbraio 2021, «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali

In accordo con le specifiche determine autorizzative dell'AIFA, la selezione del paziente da trattare con tali anticorpi monoclonali è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA e in generale ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento terapeutico. È raccomandato il trattamento nell'ambito di una struttura ospedaliera o comunque in un contesto che consenta una pronta e appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi, secondo i percorsi identificati e implementati a livello regionale. La prescrizione del trattamento deve garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza di sintomi e comunque non oltre dieci giorni dall'inizio degli stessi. La terapia con anticorpi monoclonali anti-SARS-Cov-2 dev'essere riservata, in base alle evidenze della letteratura scientifica attualmente disponibile, ai pazienti con Covid-19 di recente insorgenza, con infezione confermata da SARS-Cov-2 e definiti ad alto rischio di sviluppare forme gravi, in accordo con i provvedimenti autorizzativi dell'AIFA. Ciò premesso, passando a recenti iniziative già in corso, comunico quanto segue: è stato recentemente istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti istituzionali e professionali del mondo scientifico di elevata professionalità e competenza, inclusa AIFA, con l'obiettivo di aggiornare la menzionata circolare del del 30 novembre 2020. L'aggiornamento si sta completando alla luce delle nuove conoscenze acquisite e delle esperienze intervenute in ambito farmacologico e clinico, nonché delle recenti indicazioni dell'AIFA sui singoli trattamenti farmacologici. È comunque sempre previsto un periodico aggiornamento delle indicazioni. Si precisa inoltre che la versione aggiornata del documento sarà integrata con i tempi della terapia con anticorpi monoclonali, della gestione del paziente di età pediatrica ed evolutiva, con l'utilizzo di strumenti telemedicina e alcune specificazioni per la gestione del paziente anziano e della donna in stato di gravidanza. Le indicazioni contenute nel documento tengono conto degli studi osservazionali nazionali e internazionali e sono confermate dalle evidenze emerse dalle revisioni sistematiche della letteratura e sono conformi a quanto suggerito dalla comunità scientifica; da ultimo, tengono conto delle raccomandazioni pubblicate e divulgate dall'OMS. Dal punto di vista terapeutico, viene sottolineata la possibilità di avviare i pazienti con Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati alla terapia con anticorpi monoclonali. Inoltre, le indicazioni contenute nel documento tengono conto degli studi osservazionali nazionali e internazionali e vengono confermate dalle evidenze emerse in esito alle revisioni sistematiche della letteratura scientifica e sono conformi a quanto viene suggerito dalla comunità scientifica; da ultimo, tengono conto pubblicate e divulgate sempre dall'Organizzazione mondiale della sanità. Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnativa relativa alla nota AIFA del 9 dicembre 2020, recante i principi di gestione dei casi di Covid-19 nel *setting* domiciliare, citata nelle premesse della mozione, confermo che il TAR del Lazio, sezione Terza, con ordinanza resa in camera di consiglio il 2 marzo scorso (n. 1412 del 2021), ha accolto l'istanza cautelare e, per effetto, ha sospeso l'efficacia della stessa, fissando la trattazione nel merito il 20 2021. Atteso che l'ordinanza suddetta è stata notificata in data 8 marzo ultimo scorso ad AIFA, l'Agenzia ha tempestivamente richiesto all'Avvocatura generale di interporre appello dinanzi al Consiglio di Stato.

connesse al punto 2, che era stato dichiarato inammissibile, mi chiedevo quale fosse la valutazione. Anche le premesse, una volta votate, fanno poi parte degli atti. Il parere è negativo

Senatrice La Mura,

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica. La prossima settimana l'Assemblea si riunirà a partire da martedì 13 aprile, alle ore 16,30, per la discussione di mozioni: a firma di senatori appartenenti alla maggioranza e due a firma di senatori appartenenti all'opposizione. Le segnalazioni degli argomenti dovranno pervenire alla Presidenza entro la chiusura della seduta di domani. Le mozioni connesse per argomento, già depositate, dovranno essere indicate entro le ore 17 di lunedì 12 aprile. La ripartizione dei tempi di discussione di ciascun tema oggetto di mozioni prevede: cinque minuti per l'illustrazione e, per ciascun Gruppo, cinque minuti in discussione generale e dieci per le dichiarazioni di voto. Tendenzialmente la discussione delle mozioni sarà distribuita nel modo seguente: due mozioni martedì pomeriggio; due mercoledì mattina e due mercoledì pomeriggio. Ove i tempi non fossero sufficienti, si potrà proseguire eventualmente giovedì mattina. Altrimenti, la mattinata di giovedì 15 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni. In ogni caso, le Commissioni impegnate nell'esame dei decreti-legge pendenti al Senato sono autorizzate a convocarsi nelle fasi di discussione delle mozioni per le quali non sono previste votazioni.

relativa al Comune di San Giorgio a Cremano, nella quale abbiamo chiesto al Ministero dell'interno di attivarsi affinché venga esercitato un monitoraggio relativo alla gestione amministrativa di tale ente locale. fatto che ritengo increscioso: la Provincia di Salerno cerca restauratori gratis. Il lavoro si paga. Quello dei bandi e degli avvisi pubblici contenenti proposte di lavoro in ambito culturale da svolgere gratuitamente rappresenta un fenomeno tutto italiano che conosciamo da tempo, lesivo dei diritti dei lavoratori e di tutto il mondo della cultura, ma stavolta la Provincia di Salerno le con un avviso esplorativo, pubblicato il 26 marzo e rivolto ai restauratori, con cui realizzare uno o più progetti di restauro di opere d'arte di proprietà della Provincia di Salerno, non solo si chiede un impegno a titolo gratuito, ci si spinge anche oltre, perché in quell'avviso si può leggere testualmente che «le proposte progettuali e la realizzazione degli interventi non dovranno comportare oneri per l'ente e pertanto saranno realizzate a cura e spese del restauratore». Incredibile, ma vero. Questo episodio, signor Presidente, è la conferma di una necessaria e urgente norma sull'equo compenso dei lavoratori autonomi, infatti anche l'articolo 36 della nostra Carta costituzionale sancisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. quindi fare in modo che si riconosca pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni, impedendo che possano essere previste retribuzioni non correttamente parametrate alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste. necessario garantire il principio dell'equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi contratti con la pubblica amministrazione.

sono passati quattordici anni e non sono ancora arrivate risposte, non è cambiato nulla. In realtà sono cambiati i sindaci, i Presidenti di Regione, i Governi e i Ministri, ma nulla è cambiato per questi cittadini. Soprattutto è inammissibile

Giordano Coffen e Giovanni Borraccino, e nel conflitto a fuoco purtroppo sono stati uccisi da banditi armati con un fucile a pompa. L'assistente Borraccino rispose anche al fuoco, ma è stato

proprio in questi giorni ho voluto ricordarla all'interno di questa istituzione perché erano servitori dello Stato. Quando in una volante c'è una chiamata in radio, senti senti che la macchina accelera e ti porta a fare il tuo lavoro, senti le sirene; inizi a pensare dov'è la pistola e intervieni

ci ha portato via due servitori dello Stato. Concludo con questa frase: io, quando vedo un uomo o una donna in divisa, non mi spavento, ma mi sento sicuro. Grazie Giordano e grazie Giovanni.

al grido d'allarme e di dolore che in questi ultimi giorni e settimane da ogni parte d'Italia arriva da commercianti, imprenditori, piccoli artigiani, partite IVA e categorie produttive, cioè quella parte della società che più di altre ha pagato il prezzo delle chiusure disposte dai Governi che si sono succeduti in questo lunghissimo anno di pandemia. Le proteste di piazza delle ultime ore non sono altro che una spia di un malessere sociale profondo, che non può essere sottovalutato e nemmeno sottaciuto. Le violenze e le dimostrazioni più muscolari vanno condannate con fermezza, ma è indubbio che questo Governo questo Governo deve prendere atto che il nostro Paese ormai è allo stremo e ha bisogno di sapere quando i suoi sacrifici potranno finalmente finire e quando si potrà tornare almeno a una parvenza di normalità. Il Governo, pertanto, già dai prossimi giorni e sulla scorta dei dati epidemiologici deve iniziare a programmare le riaperture delle attività economiche. Per questo è necessario rivedere al più presto il decreto-legge che ha disposto le ultime chiusure e permettere alle attività delle aree meno esposte al contagio di riprendere il proprio sacrosanto lavoro. È questo il primo passo che va verso una ripartenza graduale, che deve completarsi nel minor tempo possibile. in tal senso le indiscrezioni secondo cui il Governo, già a partire dal 20 aprile, potrebbe considerare la possibilità di riaprire bar, ristoranti, palestre, centri estetici, esercizi commerciali e altre attività simili. Al contempo però bisogna fare di più sui sostegni alle imprese. I ristori approntati finora sono solo una goccia in quell'incendio di disagio in cui si dibattono tutti gli operatori economici. La disperazione La disperazione sociale monta sempre di più e il Parlamento e il Governo non possono far finta di niente. L'Italia deve ripartire al più presto e bisogna metterla nelle condizioni di farlo. È evidente È evidente ormai che tutti dopo un anno di *lockdown* siamo in un'altra fase e, pur tutelando la salute pubblica, adesso la priorità è scongiurare una nuova epidemia, quella economica. *(Applausi)*.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

Grazie